recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, è convertito in legge con

V. testo 2 Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

modalità diverse e nuove per gli indennizzi di questo tipo in relazione agli eventi alluvionali. Nel passato, infatti, le alluvioni davano luogo ad indennizzi soltanto con provvedimenti di protezione civile relativi alla cosiddetta fase 2, cioè quella che interviene, di regola, a maggior distanza temporale dall'evento e per importi comunque inferiori rispetto a quelli previsti dal decreto e quindi le novità consistono nella diversa gestione di questo tipo di contributo in relazione ad un'alluvione, nello stanziare importi maggiori e nella tempestività dell'erogazione. All'inizio, come ricorderà anche lei Presidente, gli indennizzi per i beni mobili non erano previsti: erano e sono previsti solo i risarcimenti dei beni immobili al 100 sebbene non fossero previsti, il fatto che l'ordinanza n. 14 del Commissario straordinario, il generale Figliuolo, desse la possibilità di caricare sulla piattaforma Sfinge anche le perizie per tali danni, faceva già presagire l'intenzione del Governo di riconoscerli in una qualche forma e così è stato e io, da romagnola, ringrazio il Governo per questa decisione che considero una decisione coraggiosa, perché credo che a nessuno sfugga il fatto che quanto previsto da questo decreto con le novità introdotte verrà a costituire un precedente che, visto il continuo susseguirsi di eventi calamitosi come appunto le alluvioni, potrebbe in futuro - anzi, sicuramente sarà così - gravare molto sulle casse dello Stato, già messe a dura prova dal superbonus e adesso forse anche dai pasticci sul reddito di cittadinanza. Quanto alla proposta di innalzare il limite massimo dell'indennizzo a 30.000 euro, fatta da una parte dell'opposizione - perché bisogna dire che su questo argomento l'opposizione si è divisa - la ritengo una richiesta decisamente demagogica e strumentale ai soli fini elettorali. Neanche l'ANCI è arrivata a chiedere tanto e ha ritenuto che 12.000 fosse già una cifra ragionevole. Non è vero che la proposta dei 30.000 euro era condivisa dalla struttura commissariale, come invece va dicendo qualche sindaco del ravennate. Capisco che in Emilia-Romagna siamo già in campagna elettorale, visto che Bonaccini è andato in Europa e a questo proposito, Presidente, mi lasci anche dire che la scelta del generale Figliuolo l'anno scorso è stata giusta, giusta, altrimenti oggi non saremmo qui per approvare una proroga di mandato, bensì per nominare un sostituto, con tutto ciò che comporta un passaggio di consegne in una fase così delicata come la ricostruzione, allora sì che avremmo sicuramente dei ritardi.

di mettere in cattiva luce il Governo solo perché è di centrodestra, solo perché, per volontà degli elettori, non è espressione del centrosinistra. Altrimenti qualcuno mi dovrebbe spiegare come mai per il sisma del 2012 in Emilia nessuno, tantomeno Bonaccini, che era (lo è ancora, non lo so) il commissario alla ricostruzione, non ha mai rivendicato indennizzi per beni mobili. beni mobili. Eppure nel caso del terremoto un precedente c'era, perché indennizzi di questo tipo furono previsti per il sisma del 2009 dal Governo Berlusconi, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3789. certo che se stessimo a quanto dichiarato dal senatore Croatti e dal senatore Manca, oggi quegli indennizzi dovremmo chiederli indietro, dovremmo chiedere di restituirli, perché a loro dire col terremoto i beni mobili non si danneggiano e pertanto tali indennizzi sarebbero stati dati impropriamente. Perché, quindi, nel 2012 non sono stati dati e oggi invece si pretendono a gran voce, rivendicando cifre importanti come fosse una prassi consolidata? Perché non si riconosce con onestà intellettuale a questo Governo il merito di aver fatto qualcosa in più rispetto a quanto era previsto l'anno scorso? Io credo che non lo si faccia perché fa comodo distrarre l'attenzione dei cittadini alluvionati; fa comodo distrarre l'attenzione l'attenzione dalle responsabilità che la Regione, che Bonaccini come commissario contro il dissesto idrogeologico, che la Schlein come assessore al Patto per il clima e alla transizione ecologica hanno avuto in questa tragedia per non avere mai fatto la dovuta prevenzione. per incapacità, per inerzia o perché la prevenzione non porta voti. Non so quale sia la risposta giusta, magari tutte e tre. Fatto sta, comunque, che la Romagna non era preparata ad affrontare l'alluvione. la costruzione delle casse di espansione era stata programmata; addirittura la cassa di espansione sul fiume Senio, che oggi è oggetto anche di un esposto in procura, già nel 2005 era considerata opera di pubblico e irrinunciabile interesse, al fine di ridurre le eventuali piene in arrivo fino a Castel Bolognese e per mettere in sicurezza i territori della bassa Romagna. Tuttavia quella cassa di espansione non è mai stata costruita e Castel Bolognese, Lugo e i Comuni della bassa Romagna sono finiti sott'acqua e ci sono state anche delle vittime. La pulizia dei fiumi non è mai stata fatta in quarant'anni; si è permesso che nei fiumi crescessero non è difficile capire che una portata dei fiumi troppo scarsa rispetto ad una piena importante può portare all'esondazione, soprattutto in pianura dove c'è una pendenza modestissima. Questo è proprio ciò che è successo a Faenza, dove ci sono state delle vittime. Per di più si è continuato a costruire sistematicamente nelle aree definite a rischio idraulico. Oggi si vorrebbe che fossero previsti anche contributi per delocalizzare quegli edifici che non sono stati danneggiati - e un emendamento in questo senso c'è ma che si trovano in zona a rischio. Sicuramente, se sarà necessario, la struttura commissariale, con ulteriori ordinanze, provvederà anche a questo; però, a parte gli edifici costruiti la domanda che bisognerebbe porsi è perché si è costruito in quelle zone a rischio. Le zone a rischio infatti, non le scopriamo solo oggi con i piani speciali; le zone a rischio ci sono sempre state, quindi sapevamo anche prima dov'erano. Oggi sentiamo il candidato della sinistra alla presidenza della Regione parlare di contrasto al dissesto idrogeologico e di azzeramento del consumo del suolo e sinceramente resto basita, perché il Comune di Ravenna è quello in Italia col maggiore incremento annuo di cementificazione. *(Applausi)*. Addirittura la prima delibera approvata dal Consiglio comunale di Ravenna dopo l'alluvione è stata la cementificazione di sette ettari di terra lungo un canale. Direi un bel cambio di rotta da parte del candidato, non c'è che dire, dire, anzi direi un performante cambio di rotta. Un'altra cosa, rispondendo sempre al senatore Manca, tramite lei, diamo un nome e un cognome a quel sindaco che, pur avendo avuto le risorse per la ricostruzione e per la messa in sicurezza del territorio, tarda nella messa a terra dei programmi e dei progetti. Quel sindaco è il sindaco di Ravenna, De Pascale, perché dei 12,3 milioni riconosciuti al Comune di Ravenna ne sono stati spesi solo… E dei 34,6 riconosciuti alla Provincia ne sono stati spesi solo… *(Commenti)*. PRESIDENTE. Senatrice, un attimo solo. Allora, colleghi, si può ovviamente dissentire sul contenuto della replica. Ho capito, ma questo, senatore Sensi, se ritiene, lei o qualcuno del suo Gruppo lo potrà far presente. *(Commenti)*. Va bene, però

mi pare di avere già risposto congruamente e assolutamente in tema. Quindi il suo intervento è assolutamente superfluo e la invito a lasciar proseguire la senatrice Farolfi. Prego, senatrice. FAROLFI, *relatrice*. Tornando agli indennizzi, l'opposizione sostiene che ci siano le risorse per innalzarli. Però io voglio fare due osservazioni. La prima è questa: è vero che nella contabilità speciale entreranno 560 milioni, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto, comprensivi dei 210 destinati agli indennizzi dei beni mobili, ma è anche vero che i rimanenti 350 è già previsto che vadano a fronte della ricostruzione privata, che deve avere la priorità. I 560 milioni infatti, insieme ai 639 che sono già nella contabilità del commissario e ai 700 messi a disposizione dalla finanziaria, concorrono ad arrivare alla cifra di 1,9 miliardi, che è proprio la cifra stimata dalla struttura commissariale per la ricostruzione privata. Fra l'altro, vorrei far notare che è una cifra molto distante dai 4 miliardi che erano stati conteggiati dalla Regione Emilia-Romagna l'anno scorso, cifra anche questa gonfiata. *(Applausi)*. La seconda osservazione - e concludo, sarò brevissima - riguarda i 210 milioni per i beni mobili. È vero che alcuni nuclei ne hanno già fatto richiesta. È vero che altri hanno già provveduto a ricomprarli usando il che - ricordo - è stato dato a 23.000 famiglie, per un totale di 103 milioni. Però è anche vero che molti la richiesta non l'hanno ancora fatta. La struttura commissariale calcola che gli aventi diritto siano 35.000 persone (nuclei familiari). Quindi noi dobbiamo dare il tempo a tutti di fare la domanda, poi magari qualcuno non la farà, perché ha provveduto in altro modo; però noi gli dobbiamo lasciare il tempo per farla. Quindi, anche se il quadro è già ben delineato, saremo in grado di capire se ci saranno dei residui solo a conclusione di tutte le procedure che sono *in itinere*, soprattutto le procedure che riguardano la ricostruzione privata, che - come ho detto prima - deve avere la priorità. Ho concluso. Grazie, Presidente.

capo di Hamas, organizzazione terroristica responsabile degli attacchi del 7 ottobre, è stato ucciso in territorio iraniano, in una situazione già maledettamente complicata dopo il vile attacco al villaggio druso, con la morte di dodici bambini, che ha portato alla reazione di Israele, uccidendo il numero due dell'ala militare di Hezbollah, il comandante Shukr. È evidente che tutto questo rischia di mettere una pietra tombale sugli accordi faticosi che si stavano raggiungendo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, proprio nei giorni scorsi a Roma. La nostra città ha ospitato l'incontro dei servizi di *intelligence* di Qatar, Egitto, Stati Uniti e Israele, per provare a trovare una soluzione. Tutto questo è saltato. Ci siamo battuti come Europa al fianco degli Stati Uniti per evitare l'*escalation*, ma oggi i rischi sono enormi. Per tale motivo chiediamo un'informativa urgente del ministro degli esteri Tajani.

all'insediamento del nuovo Presidente iraniano - e voi sapete che nel mondo islamico, nel mondo arabo e nel mondo persiano i simboli hanno un valore ancora maggiore rispetto alla nostra cultura -, rappresenta un cambio di strategia.

dalle conseguenze che questo può avere sulla geopolitica e sugli equilibri in Medio Oriente. Noi siamo, con il contingente italiano in UNIFIL, apprezzati e radicati su quel territorio da tempo, ma siamo proprio sulla linea del fronte. Uno dei possibili rischi più concreti è che la reazione sia proprio al confine del fiume Litani, dove quella che era una conflittualità a bassa intensità, che aveva portato certamente a decine di migliaia di sfollati da entrambe le parti sia in Israele che in Libano, oggi rischia di diventare il nuovo epicentro dello scontro. Hezbollah non è Hamas. Hezbollah ha un arsenale molto più sofisticato: non ha solo i razzi iraniani a corta gittata, ma ha anche gli Scud russi che possono arrivare direttamente nei Paesi arabi moderati. È evidente che questo chiede un sussulto di responsabilità da parte dell'Europa, un'azione immediata anche da parte del Governo italiano, a tutela dei nostri connazionali e anche per un'iniziativa affinché l'Europa parli con una voce sola. È evidente che, da questo punto di vista, il ministro Tajani potrà anche rispondere a un appello che è venuto da tutta la Commissione esteri e difesa ieri sulle elezioni in Venezuela, dove ancora una volta non sono stati rispettati gli standard minimi con cui si svolgono le elezioni, andando a limitare l'espressione libera del popolo venezuelano dopo tanti anni. *(Applausi)*. Da questo punto di vista, penso che ci siano tutte le condizioni per avere qui il ministro Tajani affinché dia delle risposte chiare a quest'Assemblea.

Presidente, anche noi ci uniamo alla richiesta del Partito Democratico per chiedere un'informativa urgente da parte del ministro Tajani su vicende che stanno sconquassando la la politica internazionale e che sono una minaccia per la pace non soltanto nelle regioni interessate, ma in tutto il mondo. Come è già stato detto, siamo estremamente preoccupati di quello che sta succedendo in Venezuela dove, come purtroppo era facilmente prevedibile, il regime di Maduro ancora una volta si è fatto beffe della volontà del suo stesso popolo in modo estremamente evidente, come riconosciuto dall'Organizzazione degli Stati americani e anche dai vicini del Venezuela: Paesi importanti quali il Cile e il Brasile, che hanno espresso perplessità sui dati comunicati dal Governo venezuelano e anche sulla reazione del regime di Maduro, che si sta macchiando di arresti dei principali esponenti della opposizione venezuelana. Vorremmo sentire dal ministro Tajani cosa il Governo sta facendo anche all'interno dell'Unione europea. Poi c'è il tema del Medio Oriente,

di Hamas è stato colpito da Israele proprio in coincidenza con l'attacco di Hezbollah nella parte settentrionale di Israele. Noi sappiamo che, già dal 7 ottobre, gli attacchi missilistici di droni dal sud del Libano sono stati sostanzialmente ininterrotti

che uno degli Stati che sostiene il regime di Maduro è appunto l'Iran, la stessa Repubblica islamica che sta dietro a Hezbollah, che sta dietro ad Hamas, che sta dietro agli Houthi nello Yemen. Vi è dunque un *fil rouge* che lega l'Iran, la Russia, la Cina, la Corea del Nord e che vede la loro presenza in diversi scenari e in diversi teatri della instabilità della politica internazionale. Quindi, io penso che sia fondamentale, prima della pausa estiva, che il Governo venga in Aula a informare il Parlamento su quello che sta succedendo

coinvolti in questo fenomeno di instabilità e di indebolimento delle relazioni internazionali e della pace a livello planetario. Quindi, sarebbe estremamente importante

la morte di uno dei capi militari di Hamas, che, peraltro, da quanto capisco e da quanto leggiamo sui giornali di oggi, faceva parte di una possibile delegazione in una trattativa per cercare di trovare una soluzione a quello che sta accadendo in Palestina. Capite bene, dunque, che, quando si colpisce uno di quelli con i quali si dovrebbe trattare, il rischio *escalation* evidentemente diventa ancora più clamoroso e più grande. La situazione la conosciamo tutti. Abbiamo più volte, anche in quest'Aula,

dal mio punto di vista, del Governo israeliano, che sta determinando un vero e proprio genocidio della popolazione palestinese. In conclusione, mi pare vi sia materia sufficiente per avere il Ministro degli affari esteri in Aula, di capire insieme cosa effettivamente possa fare il Governo italiano e cosa effettivamente possa fare l'Unione europea, che poi mi pare il vero grande tema di fondo di questa vicenda. Noi lo diciamo da molti mesi a questa parte. In realtà, lo dicevamo anche quando discutevamo della crisi ucraino-russa, in qualche modo denunciando un ruolo dell'Unione europea che non è sufficiente rispetto a quello che servirebbe ed una incapacità di mettere in campo una reale proposta politica. politica. Francamente, alla luce di quello che accade, mi pare sia davvero venuto il momento per provare a fare questa riflessione insieme, per cercare di capire, almeno dal nostro punto di vista, quale contributo italiano per cercare delle soluzioni che impediscano al mondo di precipitare effettivamente in una nuova guerra mondiale. Signor Presidente, come ben sa il senatore Alfieri, la Commissione affari esteri e difesa del Senato è da tempo che paventa la possibilità di un'*escalation* nella Regione mediorientale. Ne fa fede la risoluzione che abbiamo approvato all'unanimità, anche in Aula, sul conflitto israelo-palestinese, in cui tra l'altro si chiede la cessazione di ogni violenza si chiede a Israele che temperi la sua azione in risposta a quell'orrendo crimine del 7 ottobre. Insomma, la Commissione è intervenuta da subito e lo testimoniano anche le tante audizioni che abbiamo fatto, non ultima quella del Comandante UNIFIL, a cui oggi giungano i nostri sentimenti di vicinanza e sostegno per il preziosissimo lavoro che quegli uomini e quelle donne stanno compiendo dal lontano 1978 in quell'area martoriata. Vorrei fare una proposta: è evidente che la situazione oggi è gravida e il pericolo di *escalation* è ormai quasi una realtà, ma non possiamo ovviamente fermare i nostri lavori e soprattutto il nostro approfondimento su questo tema; la mia proposta è,

di Maduro di fronte alle popolazioni che vogliono esprimere e riconoscere liberamente la loro stanchezza, il loro rifiuto e sdegno verso un regime comunista che continua a opprimerle. Qual è il filo conduttore, come è stato detto? Il filo conduttore, in Medio Oriente come in Venezuela, è l'Iran, fondamentalismo iraniano che si estende e trova anche dei sostegni e degli amici in altri continenti, come in Venezuela. Ricordo - parto rapidamente da questo per poi passare a quello che sta avvenendo in Medio Oriente - la necessità di assoluta coesione e unità dei 27 Stati dell'Unione nell'affrontare la crisi in Venezuela, cosa che non è avvenuta - ricordiamoci bene - nell'autunno del 2020, quando l'Unione europea stava per adottare un sostegno esplicito al presidente Guaidó ed è stata fermata da una decisione del Governo italiano di allora di non procedere assolutamente *(Applausi)*, rompendo anche sul Venezuela, come già era avvenuto nel caso della Cina, l'unità e la coesione dell'Unione europea. Passo rapidamente a quello che avviene in Medio Oriente - e non vorrei che anche in questo delle distinzioni, delle fratture e dei giochi politici all'interno degli Stati dell'Unione - per capire esattamente cos'è avvenuto esattamente cos'è avvenuto con l'attacco che ha ucciso Haniyeh e il vice comandante degli Hezbollah, cioè ha ucciso due teste dell'idra che sono Hamas ed Hezbollah; due idre che avvolgono di aggressioni e di atrocità genocidarie lo Stato di Israele, che vogliono distruggere che vogliono distruggere lo Stato di Israele in un disegno coerente dietro il quale sta ancora una volta il regime islamico fondamentalista iraniano. È chiaro che Hamas ha una sua dimensione - come è stato detto - che non è quella di Hezbollah, che è ancora più preoccupante. Abbiamo, sul confine del Litani, una presenza italiana di un contingente di pace multilaterale

in base alle disposizioni delle Nazioni Unite non è messo in grado di controllare e di vedere le decine di migliaia di missili che sono che sono immagazzinati nelle case e sul confine. Molti di noi hanno visitato i tunnel sotterranei e le postazioni dall'altra parte del confine, dove si vede

mi riferisco a quei 12 bambini sul campo di calcio e alle decine e decine di bambini e familiari feriti da quell'attacco, che hanno subìto la conseguenza di essere minoranza in una popolazione multietnica, in un Paese democratico e civile che segue gli ordinamenti della libera democrazia, che è lo Stato di Israele. Non possiamo non esprimere solidarietà anche a queste vittime. Così come dobbiamo esprimere solidarietà alle vittime a Gaza e, poiché diciamo che il diritto umanitario a Gaza deve essere sostenuto ed applicato, non possiamo continuare a guardare solo da quella parte. Guardiamo alle vittime dello Stato di Israele dell'attacco genocidario di Hamas del 7 ottobre. Cambiamo la politica dell'Unione europea e dell'Italia nei confronti dell'Iran, dove un potere onnipotente dei militari - si chiamano Pasdaran, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica - continua a non essere sanzionato a tutto campo nelle attività economiche e strategiche, nella formazione e creazione dei droni e missili e nel portare avanti l'addestramento addirittura di reparti, come quello di Hamas, che hanno invaso Israele il 7 ottobre. Quindi, per questo credo che bisogna continuare la discussione in quest'Aula su questi temi; è un problema fondamentale di direzione della politica estera nazionale ed europea. Il prossimo Parlamento europeo è entrato in campo e deve proseguire la linea di raccontare la verità ai nostri cittadini e agire di conseguenza attraverso le istituzioni europee. *(Applausi)*.

un accordo per far uscire immediatamente un comunicato stampa a supporto della richiesta di verificare il risultato delle elezioni in maniera molto ferma.

sulla tragica e non democratica vicenda del Venezuela, dove - come abbiamo potuto osservare in queste giornate - purtroppo l'afflato democratico e il desiderio del popolo venezuelano di vedere

vigilare sul corretto svolgimento delle elezioni in Venezuela, credo sia importante fare un punto in Assemblea. Sul Medio Oriente non cambiamo la nostra posizione.

condivisibili: no ad un ribaltamento della realtà e delle responsabilità rispetto agli attacchi pesanti a cui Israele è sottoposto da molto tempo, e da parte non solo di Hamas, ma anche di Hezbollah.

apre una nuova finestra"). Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84,

Presidente, qui siamo un po' al cuore di una contraddizione che in fondo è una bugia. È stato detto che ci sarebbe stato il 100 per cento dei ristori, ma questo limite chiaramente nega quella promessa. Ora, nella storia politica del nostro Paese ci sono state tante motivazioni creative postume a promesse mancate. La più simpatica che ricordo è è del presidente Berlusconi, che disse una volta a «Porta a porta»: «Se avessi preso il 100 per cento dei voti, allora sì avrei rispettato il 100 per cento delle promesse». Qui non c'è nemmeno questa creatività. C'è una frustrazione, che giustamente le amministrazioni locali denunciano e che vivono gravemente sulla loro pelle i cittadini e le cittadine colpite da questo disastro. Signora Presidente, penso alle popolazioni alluvionate di un anno fa, che si sono viste arrivare alte personalità nei loro territori, con la promessa che non sarebbero rimasti da soli, che ci sarebbe stato un accoglimento rispetto alle loro richieste, che ci sarebbe stata un'attenzione particolare,

chiedono che vengano risarciti i danni (ad esempio, Confagricoltura Ravenna ha chiesto che i danni all'agricoltura venissero risarciti), ma non hanno ricevuto risposte; anzi, hanno ricevuto una risposta un po' piccata dalla Presidenza del Consiglio. arriva questo provvedimento, che dice: diamo riscontro a quello che avevamo promesso alle famiglie, cioè che anche gli indennizzi sui beni mobili verranno assicurati. Peccato che c'è un massimo di 6.000 euro. neanche quelle società o aziende che producono mobili che si devono montare a casa (non faccio nomi, ma tutti abbiamo capito a chi mi riferisco) fanno prezzi così bassi da ricostruire l'intero mobilio di una casa con soli 6.000 euro. Il che vuol dire che non soltanto non si dà un ristoro alle famiglie, ma che le si prende in giro, perché nessun elettrodomestico, nessun nessun elemento di mobilio costa così poco per ricostruire un intero appartamento con 6.000 euro. È passato più di un anno. Credo che quelle popolazioni abbiano dimostrato una grande dignità, rimboccandosi le maniche e andando avanti nelle proprie attività lavorative senza aiuti da parte dello Stato. Oggi ricevono uno schiaffo che forse non meritano, per la loro serietà, per la loro laboriosità e perché hanno sofferto veramente tanto e hanno visto passerelle che sono state appunto passerelle: persone straniere che nel loro dialetto dicevano di andare avanti e che non ne sarebbero stati lasciati soli. Oggi sono sbeffeggiati da un emendamento del genere. togliete il massimale di 6.000 euro e date retta agli amministratori locali, che, sentendo su di sé la responsabilità di ascoltare tutti i cittadini, a prescindere dall'orientamento politico, hanno chiesto a noi dell'opposizione (perché evidentemente la maggioranza non li ha ascoltati) di portare avanti emendamenti di dignità come questo, che non a caso è firmato da tutti i Gruppi di opposizione.

nel post-alluvione dell'Emilia-Romagna, che ha visto per la prima volta nella storia della Repubblica, su un evento calamitoso di questa specie, un intervento di 4,7 miliardi di euro, ricaduti su un territorio che ha avuto questi fenomeni alluvionali appena un anno fa. Ringrazio il Governo che, per la prima volta nella storia della Repubblica, è intervenuto subito e in tempi celeri rispetto a fenomeni alluvionali. *(Applausi)*. Lo dico perché le famiglie che erano alluvionate

E lo dico perché quelle famiglie per la prima volta riceveranno il risarcimento anche per i beni mobili: questo è un fenomeno che nei precedenti eventi calamitosi non è stato mai realizzato.

sia privata che pubblica. E quelle stesse amministrazioni locali che oggi chiedono più risarcimenti non hanno speso i soldi che il Governo ha messo a disposizione. *(Applausi)*. Sono le stesse amministrazioni locali che oggi si candidano per guidare la Regione Emilia-Romagna. Allora, se vogliamo parlare seriamente di questa alluvione e di quello che ha fatto il Governo; se vogliamo parlare seriamente dell'impegno che si sono presi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vertici

come commissario il presidente Bonaccini. Una scelta questa che si è rivelata giusta, perché poi il presidente Bonaccini ha deciso di fare altro, per cui oggi avremmo un commissario eurodeputato. Da quel giorno qualcuno ha deciso di speculare sull'alluvione. Per questo chiediamo scusa alle famiglie. L'impegno del Governo, però,

si trova ad affrontare un caso che sollecita l'opinione pubblica e che crea allarme sociale, che cosa fa? Risolve il problema? No: crea un reato. Arrivano in Commissione giustizia e ci portano un bel reato e delle belle sanzioni penali. Che cosa si fa? Si buttano all'opinione pubblica qualche manetta e un po' di tempo in galera. Lo abbiamo visto, per esempio, con il decreto Cutro: c'è un barcone che affonda, con tantissimi morti; facciamo un bel reato universale per il globo terracqueo e andiamo a prendere gli scafisti. Poi c'è la vicenda terribile di Caivano, che tutti ricordiamo, perché ha ferito la coscienza del Paese. E non vogliamo fare un bel decreto Caivano per far diventare la giustizia minorile una fattispecie che riempie le carceri, che crea sovraffollamento, che porta i ragazzi non a essere rieducati, ma ad andare a espiare la pena, così le persone saranno tranquille? a Caivano si fanno piccoli interventi, ma si fa una norma penale che va a colpire l'intero Paese, dalle Alpi fino alla Sicilia. In questo caso, che cosa succede? Per le popolazioni che sono state colpite dalle alluvioni, c'è appunto, come diceva giustamente il collega Lombardo,

lo sciacallaggio, che naturalmente è già reato e viene punito dalle norme esistenti. Questo per dire che il livello di propaganda di questo Governo è diventato completamente insopportabile. Quello che vorremmo chiedervi, signori della maggioranza, è di risolvere i problemi, cioè di andare a incidere sulle questioni che tengono in bilico e in difficoltà la vita delle persone e di non limitarvi ad agitare qualche manetta per poi, come fa qualche partito della maggioranza, dare pubblicità alle visite in carcere, che sarebbe il caso di fare prima dei decreti-legge e non dopo.

tutti i primati che il senatore Lisei ha qui vantato, questo è uno dei tanti esempi di diritti che in occasione di altre calamità sono stati riconosciuti, ma che qui non vengono riconosciuti. D'altra parte, non abbiamo ascoltato una sola risposta alla domanda se effettivamente sarebbe stato riconosciuto il 100 per cento dei danni, così come promesso all'inizio. Abbiamo dunque capito che la risposta è no. Questo emendamento è semplicemente uno dei tanti esempi nei quali il Governo è chiamato a rispettare quello che è accaduto, riconoscendo diritti che sono stati riconosciuti in passato e che qui vengono negati.

molti imprenditori sono partiti e c'è un provvedimento all'articolo 12 che è andato in questo senso, però servono più risorse e più azioni. Questo emendamento, come altri, mira proprio alla produzione agricola che

del fatto che molti imprenditori in questo momento purtroppo ancora non riescono ad attingere alle risorse che sono arrivate.

degli agricoltori e dei pescatori del nostro territorio, quindi chiedo una riflessione al Governo sull'emendamento.

mettendo in ginocchio l'intera produzione agricola della mia Regione. Ciò che mi stupisce è che, nonostante questo sia un provvedimento che parla in generale della protezione civile e che dovrebbe andare incontro alle esigenze di tutte le popolazioni

valutati i danni, quindi non c'è l'attività di valutazione di ciò che ha subìto il territorio, ritengo sia difficile che i danni siano quantificati secondo le reali esigenze. Faccio soltanto un esempio: sono stati dispersi gli alberi da frutto del territorio del Piemonte, ma anche tutta la produzione vinicola dell'alessandrino, con gravi danni per i produttori agricoli e per l'industria. un ulteriore appello affinché vengano subito erogate le risorse e non ci sia bisogno di una burocrazia che sfianca

in una situazione così drammatica, sono veramente scarse. Chiedo quindi una valutazione. Come ho detto in Commissione e ripeto in questa sede, la Regione Piemonte è governata dal centrodestra, quindi non ci dovrebbe neanche essere quell'accanimento "terapeutico" contrario che avviene in Emilia-Romagna in quanto Regione non amica.

che le popolazioni del Piemonte hanno subito nei mesi scorsi.

il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo, a mio avviso, mostra tutta la confusione che regna nella maggioranza maggioranza e che, secondo me, si salda con un'improvvisazione totale. Io francamente non comprendo le ragioni per le quali si possa esprimere un parere contrario su un emendamento che, di fatto,

un ottimismo da parte del senatore Lisei sull'azione del Governo, ritengo che non approvare questo emendamento sia un'ammissione di colpa e la dimostrazione che questo Governo fallisce nella ricostruzione. infatti strade sulle frane e ripristinare immobili nelle immediate vicinanze dei corsi d'acqua non corrisponde all'attuazione di un piano straordinario per l'adattamento ai cambiamenti climatici, dimostra che avete come idea esclusivamente quella dell'emergenza e della ricostruzione di opere di somma urgenza senza una visione strutturale del futuro del nostro Paese senza avere nella testa l'idea che i cambiamenti climatici ci appartengono e richiedono misure straordinarie per fare prevenzione. Come si fa ad esprimere un parere contrario su questo emendamento? lo ribadisco - che dietro a questa ricostruzione ci sia la politicizzazione di uno scontro tra i diversi livelli istituzionali, che si rivelerà un danno per il Governo e per il Paese. Provate a ripensare alle cose che state dicendo e ai pareri che state affrettando; se volete che la ricostruzione funzioni, il commissario dev'essere rapidamente nelle condizioni di approvare e periziare gli immobili che non sono collocati in zona congrua. Se vogliamo fare un qualcosa di utile per le future generazioni e non per la vostra propaganda, cambiate strada e cambiate idea; provate a ricostruire una relazione proficua e positiva con i livelli delle Istituzioni, che non si governano con dei capibastone e con dei capipartito,

non di merito. Su un emendamento di merito, si risponde in termini di merito. State facendo solo propaganda, altro che

che questo Governo aveva promesso di ricostituire, approvando un ordine del giorno, che siamo ancora in attesa che si concretizzi. Nel frattempo, c'è la possibilità di costruire interi territori, riparando, ripartendo ed evitando gli errori fatti nel passato, eppure abbiamo un parere negativo su un emendamento molto semplice.

un emendamento che riguarda gli avvalimenti: la copertura economica sulle convenzioni, sia con le amministrazioni sia con le società, è dentro il 2023; con questo emendamento chiediamo di arrivare a garantire continuità al 2024 solamente per fare una programmazione dei lavori delle aziende.

affrontare questo momento difficile per quanto riguarda le nomine di dirigenti, utilizzando quelli selezionati dal progetto «Mille esperti PNRR». La maggior parte delle questioni di cui parliamo adesso riguarda le difficoltà dei sindaci sul territorio e l'assunzione dei dirigenti è fondamentale in questo momento, quindi c'è bisogno di dar loro manforte con strumenti operativi. Pertanto, se potete capire l'entità della difficoltà degli amministratori in questo momento, diamo loro dei dirigenti per poter affrontare in maniera seria questo passaggio.

queste attività sono assolutamente indispensabili per qualsiasi pianificazione. Investire in questo progetto significa accelerare i processi di pianificazione per rispondere ai problemi del dissesto idrogeologico, ma anche sismico. Il Governo Conte ha investito 11 miliardi in due anni su questo progetto. questo progetto. Questo Governo non ha capito l'importanza di investire nella CARG, ma l'emendamento in esame spinge il Governo a farlo, perché prevenire è meglio che curare. Se però non investiamo negli strumenti che ci consentono di prevenire, non stiamo facendo un buon lavoro e un buon servizio al Paese e ai cittadini.

vorrei chiedere al Governo e al relatore un ripensamento rispetto al parere contrario su questo emendamento, che mira a semplificare la vita a Comuni che hanno avuto aggravi burocratici molto forti in questi ultimi mesi e che rischiano, per meri problemi formali, di perdere l'accesso a finanziamenti importanti. Non vedo per quale ragione si sia adottata una linea di contrarietà a questa richiesta, che è elementare e di buonsenso. È molto triste quando anche il buonsenso diventa difficile da raggiungere. Mi appello al Governo e alla relatrice per una diversa valutazione di questa proposta emendativa.

aveva la contrarietà del MEF per ragioni di bilancio, ma non si capisce, non lo abbiamo capito e non ci è stato spiegato per quale motivo una proroga dei termini determini problemi di bilancio. È diventato un intercalare e il Governo nega anche richieste ragionevoli che vengono dalla maggioranza.

il senatore Fina mi segnala che è saltata, per un disguido, la mia firma, che vorrei aggiungere, a questo emendamento.

appaiono del tutto inadeguate a far fronte a tali legittime aspettative.

la crisi idrica nelle due principali isole italiane, la Sicilia e la Sardegna, anche se sappiamo che è un tema che riguarda tutto il Sud. Qui non c'è stata occasione di portarlo avanti, ma è un tema sul quale diciamo è importante impegnarsi tutti. Le risorse che fino ad oggi sono state stanziate complessivamente sono inferiori ai 40 milioni. A fronte di questo abbiamo dei danni che, secondo la Lega delle cooperative, ieri già superavano i quattro miliardi. La proposta che noi facciamo qui è quella di utilizzare i fondi sviluppo e coesione per iniziare a dare una effettività ai progetti che sono stati realizzati. Ci sono ventotto interventi, ma pochissime risorse fino adesso impegnate.

Naturalmente, non pretendiamo che questa sia la soluzione a tutto, ma in un decreto che si occupa del post-calamità e di protezione civile non ci poteva non essere una parte riguardante l'emergenza e la siccità.

di votare favorevolmente a questo emendamento che interviene per riconoscere la crisi che sta colpendo, per via della siccità, il comparto agricolo, in particolare quello dei lavoratori a tempo determinato che non hanno alcun ristoro

stabilendo che la Fondazione Milano Cortina 2026 opera in regime di diritto privato, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e non riveste la qualifica di organismo pubblico. A parte il fatto che le società pubbliche operano in regime di diritto privato ma mantengono la natura pubblica, faccio presente che questa interpretazione va in contrasto con la direttiva europea n. 24 del 2014, che è stata recepita anche da diverse sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Cassazione a sezioni Unite con sentenze del 2021 e del 2023.

Faccio anche presente che la situazione economica e il bilancio di questa società sono fortemente in rosso, con un debito al 2023 di 101 milioni

una nuova finestra"). Informo che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata per le ore 15,45. Per l'espressione dei pareri sui tre emendamenti mancanti servono ancora dieci minuti alla Commissione bilancio.

«*Nel capo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-bis. - (Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,

della legge 23 dicembre 2014 n. 190, relative al sisma del 1990*) 1. Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è istituito, trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Ragusa. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

alinea, è stabilita la data di soppressione della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Fino alla data indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2024, detta Struttura di supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso di cui al comma 13, lettera ultimo periodo, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza periodica, almeno mensile, apposita relazione al Commissario straordinario di cui al comma 1, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

dei Capigruppo ha stabilito che, nella seduta di oggi, dopo la votazione finale del decreto-legge in materia di ricostruzione e protezione civile, si passerà all'esame del disegno di legge per la proroga del termine di adozione di testi unici in materia tributaria. La seduta di domani, con inizio alle ore 9, prevede la discussione del decreto-legge in materia penitenziaria e di giustizia civile e penale. Il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento al termine della discussione generale. Pertanto la Conferenza dei Capigruppo ha organizzato il relativo dibattito, stabilendo di passare alle dichiarazioni di voto e alla chiama. Restano confermati gli altri argomenti già previsti nel calendario dei lavori. La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi lunedì 5 agosto.

oggi in Aula siamo chiamati ad esprimerci su un provvedimento di ampio respiro, con una visione strategica. È un testo che si pone l'obiettivo di ricostruire il tessuto prima sociale e poi economico delle città e delle aree ferite da eventi calamitosi. Far tornare a vivere quei luoghi è un dovere, far tornare a battere il cuore di quei luoghi è un obbligo morale: è la sola risposta alla morte, al dolore e alle ferite che altrimenti rischiano di spegnere le luci di quei campanili, di quei borghi e di quelle città che rappresentano il tessuto della nostra Italia. Ricostruire e mettere in sicurezza, riconnettere delle aree e riallacciare i rapporti è l'unica strada per dare risposta a quei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, Regioni che lo scorso anno sono state interessate da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità, che hanno provocato gravi danni alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati e alla rete dei servizi essenziali e idraulici. Grazie all'accurato lavoro svolto dal Governo Meloni, in particolare dal ministro Nello Musumeci, e a quello in corso di svolgimento in Parlamento, a breve l'Italia farà tutto questo. La nostra Nazione potrà dotarsi di una legge in materia di ricostruzione post-calamità che comprende un *corpus* di norme in grado di garantire maggiore programmazione, omogeneità ed efficacia degli interventi. Si tratta di una pietra angolare e di un modello nuovo per rispondere alle emergenze e poi passare alla fase di ricostruzione, un passo in avanti deciso per il nostro Paese. Riconosciamo dei contributi a soggetti privati titolari di immobili che abbiano che abbiano subito danni a causa di un evento calamitoso. Per questo stanziamo oltre 550 milioni ed un massimo di 6.000 euro per abitazione: è un qualcosa che non è mai stato fatto negli anni precedenti e in eventi di questo genere. Allo stesso tempo, l'articolo 2 è volto ad accelerare le procedure di ristoro nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata per garantire quanto prima il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni. Al fine di promuovere la sicurezza del territorio e della popolazione delle aree maggiormente colpite dall'evento alluvionale, liberando al contempo le aree a maggior pericolosità idrogeologica, anche a seguito degli studi preliminari del Piano speciale sul dissesto, prevediamo la possibilità, per le imprese e i cittadini, di acquistare aree alternative o immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei Comuni in cui è ubicato l'immobile privato danneggiato. La proroga dell'incarico del commissario per la ricostruzione risponde a un'evidente esigenza di continuità sugli interventi e garantirà un'attenta attività ispettiva, di controllo, vigilanza e repressione dei potenziali illeciti collegati all'utilizzo dei conti pubblici. Per assicurare continuità nei controlli, le azioni di verifica saranno a cadenza mensile: è la dimostrazione che non sarà lasciato spazio al caso. Le opere andranno realizzate nel perimetro della legalità ed effettuate a regola d'arte. In caso di accertamento di illeciti, le somme recuperate non andranno perse, ma saranno riversate in un apposito capitolo, per una successiva per una successiva riassegnazione a territori colpiti dalle alluvioni a partire dal maggio dello scorso anno. In questo percorso non lasciamo soli i Comuni: il loro ruolo sarà determinante nella ricostruzione e sarà centrale vestiranno i panni dell'organo intermedio. Gli enti locali, i sindaci e gli amministratori sono donne e uomini in trincea, in prima linea: sono loro che hanno il compito di continuare a erogare i servizi, allo stesso tempo collaborando a mettere a terra tutti gli interventi di ricostruzione progettati. Possono farlo con una struttura adeguata. Per questo, attraverso il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge, prevediamo la possibilità per gli enti locali di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi per assumere profili professionali indispensabili per raggiungere in breve tempo questi obiettivi. Per procedere con celerità, ampliamo la platea dei soggetti attuatori, pianificando specifiche convenzioni per gli interventi previsti, soprattutto per velocizzarli. Riconnettere il tessuto sociale è un obiettivo che si può raggiungere solo attraverso la ricostruzione della rete infrastrutturale e viaria. Infatti, con l'articolo 7 rispondiamo all'esigenza di operare soprattutto nelle fasce di territorio collinari e montane, attraverso soggetti di comprovata esperienza nel settore ingegneristico. In questo sarà determinante anche la capacità progettuale del gruppo Ferrovie dello Stato, anche in considerazione del fatto che i fenomeni di dissesto hanno interessato strutture del gruppo ferroviario, con uno stanziamento di oltre 250 milioni. Anche all'ANAS sarà data la possibilità, attraverso le proprie capacità progettuali ed esecutive, di intervenire in maniera efficace e dando sostegno alle amministrazioni locali e ai piccoli Comuni montani (in difficoltà soprattutto per carenze di personale formato formato e attento a situazioni di questo genere, che magari non hanno mai vissuto in passato) che più di altri hanno bisogno di non essere lasciati da soli. Con il piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali non tralasceremo gli interventi sulle opere di urbanizzazione primaria, come il collettamento collettamento fognario e per un piano speciale per i beni culturali, anche per rilanciare il turismo in alcune aree colpite negli anni precedenti. Ci sarà un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite e sarà data priorità alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, perché solo ripopolando i territori possiamo sul serio contrastare il rischio idrogeologico. È innegabile che l'abbandono delle aree, la mancanza di cura, attenzione e manutenzione genera e può generare simili drammi. altro aspetto riguarda lo stato di emergenza e il suo superamento con le attività di protezione civile. Attraverso l'articolo 8 estendiamo l'autorizzazione alla spesa di 92 milioni di euro per il 2023 e di ulteriori 50 milioni annui dal 2024 al 2027.

di Brindisi, garantendo la sicurezza dei più grandi Capi di Stato internazionali. L'Italia è un territorio bellissimo e allo stesso tempo fragile. I Campi Flegrei rappresentano in pieno questa sintesi: uno dei vulcani più pericolosi e complessi al mondo, un'area che purtroppo, nonostante i pericoli incombenti, ha visto uno sviluppo irragionevole. È inutile nascondersi e negarlo: chi doveva vigilare non lo ha fatto. Il Governo Meloni interviene nell'immediato per dare risposte ai cittadini e superare l'emergenza. Per la riqualificazione sismica e il ripristino degli edifici residenziali inagibili si riconosce un contributo per gli interventi di ripristino in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dopo il sisma del 20 maggio 2024. Il nostro è un Paese caratterizzato da un'accentuata vulnerabilità sismica ed idrogeologica, che non hanno pari a livello europeo. In Italia ci sono 678.000 frane attive, due terzi di tutta l'Europa. Questa nostra fragilità rischia di essere accentuata dall'avanzare della crisi climatica, dal momento che l'abbandono delle aree interne e l'assenza dell'uomo determinano un ampliamento della portata di eventi catastrofali. Dunque dobbiamo essere consapevoli del fatto che crisi demografica e crisi climatica sono due facce della stessa medaglia e che di ciò dobbiamo tener conto nell'ambito del processo di ricostruzione, che è una creatura viva e in costante evoluzione. Come sottolineato dal ministro Musumeci (è bene ricordarlo anche qui), la ricostruzione deve essere un'occasione di prevenzione, di ricostruire meglio e di innovazione. Il motto "dov'era com'era" ci porta lontani dal rendere i nostri luoghi più abitabili. Abbiamo a disposizione nuove tecnologie, la digitalizzazione, ed è dunque necessario farne buon uso. È per questi motivi e per altri che il nostro Gruppo darà il voto favorevole alla conversione di questo decreto-legge.

quello che dopo un anno e mezzo non potete più fare è dire che tutte le responsabilità esistenti sulla faccia della terra dipendono dai Governi precedenti e non dal vostro, perché, dopo un anno e mezzo, non dico tanto la responsabilità, ma la visione di dove volete portare il Paese deve essere quantomeno tracciata, posto che due partiti su tre della vostra maggioranza già hanno governato negli anni precedenti. *(Applausi)*. Accusare le forze politiche dell'opposizione di non aver fatto mai prevenzione, in un provvedimento che parla del post-calamità, di protezione civile e di eventi internazionali sportivi (su tutti Milano Cortina), non è ingeneroso: è falso. È falso perché chi le parla orgogliosamente rivendica due misure del Governo Renzi: Casa Italia, per la ricostruzione del post-terremoto dell'Italia centrale,

E allora, se questo è il provvedimento che dà la visione di questo Governo, che è il primo Governo politico - come lo definite voi - dopo molti anni, si tratta di una visione altamente insufficiente. Lo è perché non c'è la prevenzione, innanzitutto; avete bocciato tutti gli emendamenti che riguardavano la prevenzione. Lo è perché, se deve essere un decreto che dà dei ristori a chi ha subito un danno, si tratta di ristori *spot*, non c'è un criterio oggettivo. Non lo dicono soltanto le forze politiche, ma banalmente i cittadini dell'Emilia-Romagna. Forse sono diventati tutti diventati tutti di sinistra; ma, visto che ho avuto la fortuna di essere eletta in quel territorio, mi ricordo che il partito di Fratelli d'Italia era il secondo partito, con pochi punti percentuali di distacco dal Partito Democratico. Ciò vuol dire che, in questi anni, anche chi vi ha votato è rimasto profondamente deluso da come è stata gestita l'emergenza post-alluvione. Avete nominato un commissario che non era politico. Voi che vi vantate così tanto di voler far tornare all'onere della parola politica quel significato importante, avete scelto un commissario tecnico, ma non gli avete dato le risorse e soprattutto

tanto è vero che ha messo delle proprie risorse per ricominciare a creare prodotto interno lordo non soltanto per quella regione, ma per il Paese. Non ha però avuto soddisfazione e cito in particolare gli agricoltori di Ravenna. Sono passati da essere eroi ad essere dimenticati nel giro di poche settimane; eroi perché l'acqua non stava per entrare nei loro campi *(Applausi)*, ma hanno scelto loro di tutelare il patrimonio dell'Unesco, cioè le bellezze monumentali che sarebbero state devastate dall'acqua e dal Hanno ricevuto gli applausi, ma non hanno ricevuto le risorse; e quando si sono permessi di dirlo, avete bacchettato l'associazione agricola di cui fanno parte, dicendo che quell'associazione attaccava politicamente il Governo. Come se dire di non aver ricevuto risorse sia una critica politica.

ridimensionando le aree incluse nella zona rossa, quella più sensibile, nel momento in cui ogni tre per due ci sono scosse telluriche ed emergenze dovute al fatto che non c'è la fine

scagliato contro l'abusivismo e abbia fatto provvedimenti per abbattere tutti gli ecomostri della sua Regione. Quindi trovo veramente che lo scaricabarile non abbia sortito un buon effetto e non sia stato particolarmente elegante.

Quando ho letto la norma che prevede un soggetto privato per meglio spendere le risorse pubbliche mi è venuto da sorridere, perché mi sono ricordata a un certo punto che nella mia Commissione abbiamo analizzato anche il

avevano bisogno, anche dopo il blocco del superbonus, di avere uno strumento normativo per poter accedere a norme più semplici per procedere nei lavori, ma si sono viste di fatto bloccare intere gare d'appalto. Questo è un provvedimento che non ci convince perché non dà le risposte che servono né a chi ha subito un danno né a un Paese che deve profondamente cambiare. Arriva dopo il salva casa di Salvini un provvedimento dove si dice che si è contro l'abusivismo edilizio e c'è un Ministro che si scaglia contro quei Comuni intorno al Vesuvio che, secondo lui, hanno il primato dell'abusivismo: mi viene abbastanza da sorridere. Evidentemente i due Ministri non si sono parlati quantomeno quando hanno dovuto rilasciare dichiarazioni pubbliche, perché sembra veramente una presa in giro e non serve a Milano Cortina. Concludo proprio con riferimento alle Olimpiadi. A me dispiace molto che il Comune di Torino all'epoca abbia abbandonato il progetto olimpico. Mi dispiace, perché avevamo le infrastrutture Poi, dopo che è arrivato il nuovo sindaco Lo Russo e con il presidente della Regione Cirio, sia il Comune di Torino che la regione Piemonte hanno cercato di rientrare nella corsa olimpica, un po' rimbalzati. Sono contenta che, per le Olimpiadi del 2030, la Francia sceglierà Torino, utilizzando l'Oval per il pattinaggio. Sono molto rammaricata che questa scelta non l'abbia fatta Milano, preferendo costruire un altro palazzetto dello sport; o Cortina, preferendo sradicare altri alberi piuttosto che utilizzare la pista del bob di Cesana Torinese. Mi dispiace,

Presidente, anche per ragioni di tempo io affronterò soltanto un punto di questo decreto, quello che riguarda i Campi Flegrei. contro il provvedimento: con un certo rammarico, non lo nego. Lo faremo, però, perché questo decreto affronta, dal nostro punto di vista, in maniera insufficiente quella che invece è una enorme vicenda, che riguarda peraltro centinaia di migliaia di persone, e sulla quale ci si sarebbe attesi uno sforzo vero da parte del Governo, con un lavoro magari unitario tra Stato centrale, enti locali, comunità,

ma è a mio avviso molto grave la speculazione politica vera e propria di cui il ministro Musumeci in particolare, che mi dispiace oggi non ci sia, si è fatto portatore in tutti questi mesi. Io considero totalmente insopportabile, come è stato ricordato anche da altri colleghi, scaricare le responsabilità sui sindaci del territorio, come se fossero colpevoli di non aver fatto abbastanza per ridurre la pressione abitativa. Tra l'altro, è stato ricordato ieri dalla senatrice Valente che fu proprio il centrodestra ad osteggiare la legge regionale campana del 2003, che si poneva esattamente l'obiettivo di ridurre la pressione abitativa nelle aree più a rischio. Insomma, siete stati i campioni dei condoni edilizi e del consumo di suolo: veramente, ci manca solo questa speculazione politica insopportabile. Basta propaganda. Basta, una volta per tutte. *(Applausi)*. Servono, invece, fatti concreti e risposte: a partire, per esempio, dalla questione enorme delle famiglie sfollate a seguito delle diffide di agibilità o agli ordini di sgombero. Famiglie che devono essere messe nelle condizioni di tornare nelle proprie case in tempi ragionevoli. Si tratta di oltre 1.500 persone che sono in una condizione estremamente precaria, per essere gentili, alle quali il il Governo si limita soltanto ad assicurare, per un tempo limitato, un contributo all'affitto. Contributo che, nella grande maggioranza dei casi, si rivelerà purtroppo insufficiente per coprire i costi ormai altissimi delle locazioni private. Si sarebbero dovute investire risorse considerevoli nel recupero degli edifici privati e pubblici, danneggiati in particolare dall'ultima scossa più grave, quella del 20 maggio. E i costi dei lavori per la messa in sicurezza non possono certo ricadere sui singoli proprietari, come se si trattasse di un loro normale obbligo di manutenzione. Si investono 20 milioni per il 2024 e 15 milioni per il 2025 e 2026 negli interventi di riqualificazione sismica e per la riparazione dei danni delle case sgomberate e dichiarate inagibili. Sono cifre, però, lo capite bene, totalmente insufficienti rispetto alle reali esigenze. Dei 420 milioni diluiti sino al 2029, previsti per gli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e per le infrastrutture di trasporti e servizi, la metà sono detratti dal fondo sviluppo e coesione della Regione Campania. Il tutto peraltro condito dal solito ricorso al commissariamento, che non si capisce bene cosa potrà fare senza risorse disponibili. In realtà, credo che anche questa del commissariamento sia una scelta molto discutibile, non solo perché abbiamo già la legge speciale n. 189 del 1984 con un commissario, legge che fu dovuta alla crisi bradisismica dei primi anni Ottanta e che è stata un totale fallimento, perché non ha previsto un concessionario unico per le vie di fuga, che ancora oggi non sono state completate, ma anche perché più che un commissario servirebbe una cabina di regia composta da tutti gli enti coinvolti per evitare, per esempio, che su un tema grande come quello della pianificazione urbanistica venga sottratta la competenza alle istituzioni democraticamente elette nei territori. Tutto questo, peraltro, senza che sia stato mai dichiarato alcuno stato di emergenza nazionale per i Campi Flegrei e senza che siano state impegnate le risorse necessarie per intervenire con azioni risolutive. In queste condizioni, nelle modalità indicate dal decreto-legge e con le scarse risorse messe in campo, al commissario altro non spetterà che magari decidere qualche consulenza, ma non certo quella di programmare interventi o opere infrastrutturali. Noi crediamo, Presidente, che esiste un solo modo per rendere tollerabile la convivenza della comunità con il bradisismo, perché alla fine di questo si tratta: intervenire su tutti gli edifici per renderli sicuri e antisismici, in grado cioè di sopportare eventi di magnitudo di lieve o media entità. Occorrerebbero controlli veloci, certificazioni sulle condizioni dei fabbricati, in modo da quantificare le risorse necessarie per salvaguardare il patrimonio abitativo e anche, naturalmente, il tessuto sociale esistente. I paesi ricompresi nella zona bradisismica vanno difesi nella loro totalità, che è fatta di case, ma è fatta anche di scuole, di chiese, di pubblici esercizi, di luoghi di socializzazione e quindi di persone, di residenti, di lavoratori, di cittadini, di rapporti umani, di legami e di identità, risorse che andrebbero concentrate per l'appunto nella messa in sicurezza degli edifici, senza alimentare nuovi cantieri decennali o pozzi senza fondo, come purtroppo succede troppo spesso. garantiti i diritti, a cominciare dalla salute: le prestazioni sanitarie pubbliche, per esempio, non possono essere ridimensionate in nessun caso diverso dal preallarme per rischio vulcanico di allerta arancione. Insomma, questi territori hanno bisogno di una concreta prospettiva di rinascita. Non si può rinunciare allo sviluppo, che nei Campi Flegrei vuol dire il porto, la tutela delle attività produttive, le attività tradizionali del mare e del commercio e vuol dire anche turismo culturale. Su questo vorrei vorrei fare un'ulteriore considerazione finale: trovo davvero molto discutibile che nel decreto non compaia mai la parola «archeologia» e nemmeno la previsione di un fondo dedicato ai beni culturali. Lo trovo assurdo, anche perché parliamo - lo dico ai colleghi che magari lo sanno di meno - di un territorio ricchissimo di beni archeologici, che, in larga parte peraltro, ricadono nelle proprietà private in zona rossa. Invece, non si prevede nulla per il patrimonio; il Ministero della cultura ha censito i beni culturali in consegna allo Stato nella zona rossa, ma non ha preso in considerazione i tantissimi beni archeologici dei privati. Infine, su un'altra questione molto rilevante, quella del Rione Terra e del Parco archeologico, vorrei ricordare che i cittadini, in particolare di Pozzuoli, che è il Comune dove queste aree incidono, sono già stati privati in passato di un luogo dal fortissimo valore identitario per la comunità locale, che fu acquisito dal Comune e poi però destinato ad alberghi di lusso. Fortunatamente, nei trent'anni successivi, con i finanziamenti della Regione Campania, il Rione Terra è stato restituito al pubblico, è diventato una straordinaria realtà archeologica del territorio. Ecco, il solo fatto che questo decreto-legge non preveda nulla sul tema della fruibilità di questi patrimoni archeologici, attorno ai quali ruota tutto il sistema degli operatori dei beni culturali, penso che la dica davvero lunga sulla miopia del Governo e sulla sua incapacità di soddisfare le attese del territorio. Peraltro, lo vorrei davvero ricordare, stiamo parlando di un luogo - Pozzuoli, l'antica Puteoli - che ha una storia straordinaria, cominciata, pensate voi, nel 194 avanti Cristo, una storia che va avanti ancora oggi; la storia di quella che fu nell'antichità una città città straordinaria, cosmopolita e multiculturale; una storia, un patrimonio culturale, quindi, che ha un enorme valore identitario e che bisognerebbe rispettare molto assieme, ovviamente, a tutti quelli che a Pozzuoli ci vivono ancora oggi. anche per queste ragioni e naturalmente per tutte quelle che sono state ricordate in discussione generale dalla mia collega Floridia, noi di Alleanza Verdi-Sinistra voteremo convintamente contro il decreto-legge

non erano critiche - lo dico da responsabile nazionale del settore casa del mio partito - ma erano osservazioni sul fatto

la maggioranza è pronta a intervenire. Veniamo al decreto-legge in esame: oggi esaminiamo due interventi urgenti emanati a circa un mese di distanza per far fronte alle conseguenze di due eventi naturali nefasti: il primo prevede la ricostruzione post-alluvione, il secondo riguarda i rischi del bradisismo. L'occasione è anche utile per introdurre disposizioni più puntuali in tema di protezione civile. Per quanto riguarda le alluvioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, è stata prevista una maggiore semplificazione per accedere ai contributi. Inoltre sono state implementate norme che consentono ulteriori assunzioni nella pubblica amministrazione, oltre a nuove disposizioni per contrastare il dissesto idrologico-ferroviario. Il decreto ridisegna la contribuzione pubblica nelle tre Regioni coinvolte dall'alluvione dello scorso anno. I contributi previsti possono essere destinati al rimborso fino al 100 per cento delle spese occorrenti per l'acquisto di aree edificabili alternative o di immobili immediatamente disponibili per destinazione residenziale o produttiva nello stesso Comune del bene danneggiato. Il commissario straordinario potrà avvalersi di enti pubblici e organi statali per effettuare le verifiche sugli interventi per i quali siano stati concessi i contributi per la ricostruzione. Per le assunzioni a tempo determinato negli enti locali è prevista la facoltà di attingere anche alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni. Sempre il commissario straordinario e la società RFI sottoscriveranno un'apposita convenzione per attuare interventi sulla rete ferroviaria per risolvere i problemi del dissesto idrogeologico lungo le infrastrutture dedicate ai treni. Viene estesa la copertura dei contributi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in calamitosi verificatisi nel 2022 e 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e per i quali non siano già stati previsti finanziamenti. A differenza dell'altra parte del decreto-legge, che si occupa di guarire le ferite dell'alluvione, con le norme ora qui trasfuse dal decreto Campi Flegrei si punta alla prevenzione dei danni in una zona soggetta ad attività di bradisismo.

L'obiettivo è la tutela e la riqualificazione del patrimonio edilizio, sia pubblico che privato, oltre agli interventi per le infrastrutture dei trasporti e dei servizi essenziali. Per realizzare questi obiettivi viene individuata la figura del commissario straordinario per l'attuazione del PNRR in quest'area, che resterà in carica fino al 2027. Il commissario potrà adottare misure di accelerazione dei lavori anche in deroga, inserendo nel programma di riqualificazione anche varianti agli strumenti urbanistici, in modo tale da semplificare le procedure e accelerare una macchina amministrativa ferma che deve essere più efficiente. Sono infatti necessari interventi urgenti, soprattutto per spendere in modo appropriato le risorse già assegnate. La stessa logica guida la volontà di intervenire sulla mobilità e per garantire la continuità scolastica negli edifici, ad esempio, di Pozzuoli, che sono stati danneggiati e sgomberati perché inagibili. Inoltre, ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità, viene riconosciuto un contributo per trovare una sistemazione autonoma. La disposizione a nostro giudizio più importante è quella che pone le basi strutturali per poter convivere con il fenomeno del bradisismo in maniera sicura, stabilendo specifici divieti in relazione al rilascio dei nuovi titoli edilizi per interventi di nuova costruzione, inoltre un elenco degli edifici privati che abbiano una vulnerabilità sismica nei comuni interessati. In tutti questi casi si prevedono interventi di riqualificazione edilizia anche con procedure dedicate e appositi contributi alle famiglie. Sotto il profilo finanziario il decreto Campi Flegrei mette in campo circa 400 milioni di euro. Voglio ricordare che per le alluvioni del 2023 il Governo con più provvedimenti ha messo in campo più di 6 miliardi di euro. in sintesi, di misure concrete per porre rimedio all'azione nefasta delle forze della natura - l'alluvione e il bradisismo - spesso agevolate dalla precedente incuria dell'uomo. Come ho avuto modo di dire in precedenti interventi, purtroppo io sono un "alluvionato" del 1994 (l'alluvione del Piemonte) e so bene quali siano le esigenze di chi viene colpito da queste tragedie. So bene cosa vuol dire sentirsi il fango addosso anche dopo che ti sei lavato decine di volte. Conosco quel suono che continua a riempire le orecchie e l'acqua che ribolle insinuandosi nella tua casa. Ricordo l'angoscia di quando guardavo fuori dalla finestra e, nel buio totale, vedevo sagome che galleggiavano e pregavo che non fossero persone, amici, parenti. Per questo posso dire che con una serie di decreti mirati dedicati alle popolazioni coinvolte nei disastri naturali di questi anni, il Governo si è dimostrato attento ai bisogni dei cittadini colpiti da eventi che hanno cambiato improvvisamente e forzosamente il corso della loro vita. Un Governo che sta lavorando per restituire la normalità della vita a chi vuole solo una vita normale. Un Governo così è un buon Governo e merita il nostro sostegno.

e colleghe, membri del Governo, grazie alla vostra spiccata capacità di sintesi oggi, visto che siamo ancora in tempi di saldi, mostrandovi sempre sul pezzo, siamo in Aula qui a votare ben due decreti-legge in uno; della serie due per uno. La votazione di questo provvedimento arriva dopo settimane di indiscutibili successi, sia a livello nazionale che internazionale, culminate con la letterina a Babbo Natale che la *premier* Meloni ha inviato a Ursula von der Leyen. quanto siamo lontani da quei tempi in cui si usava ripetere che con Giorgia in Europa era finita la pacchia! Quanto siamo lontani da questa frase che, con il consueto *aplomb* istituzionale, la Presidente rivolgeva alle istituzioni comunitarie, rivelando sin da quello che sarebbe stato un approccio fallimentare su tutta la linea e che non ha fatto altro che mettere in evidenza la vostra totale incapacità e inconsistenza. Le vostre trasformazioni sono innegabili e sotto gli occhi di tutti, come quella di un Vice *Premier*, per esempio, che si sente un tantino sotto assedio. Qualcuno gli ha rubato voti e anche la scena e quindi cerca di spostarsi un po' più a destra ed è passato con molta *nonchalance* dall'affidarsi dall'affidarsi al cuore immacolato di Maria ad un più terreno generale di fanteria, pur di restare a galla, ma questo di certo non permette ai treni di arrivare in orario, ma che fa? Tanto lui pensa solo a una cosa: al Ponte

che negli anni passati non c'è mai stata una programmazione seria della crisi idrica. Ebbene, siamo qui a ricordarle che negli anni passati, esattamente dal 2017 al 2022, è stato lei il Presidente della Regione Sicilia. *(Applausi)*. meno male che ci siamo noi a ricordarvi di queste cose. Questo provvedimento, al pari degli altri che state portando in Parlamento, è solo un'altra pagina mal scritta dei vostri fallimenti. Le misure sono inadeguate e insufficienti, abbiamo provato ad aggiustare il tiro in Commissione, ma come al solito avete deciso di andare dritti per la vostra strada. In Commissione abbiamo toccato con mano l'inconsistenza di questo Governo e al contempo abbiamo sentito dichiarazioni da parte di parlamentari della maggioranza che dicevano che è la prima volta che un Governo stanzia dei soldi per l'acquisto di mobili danneggiati. Eh già, complimenti per la fantasia, torno a dire. Peccato che i 6.000 euro ad abitazione che avete promesso siano solo una goccia nel mare rispetto alle spese che si trovano ancora ad affrontare

sua, ministro Musumeci, rientri nella cifra di 3.200 euro, oppure se la vostra camera da letto o la cameretta dei vostri figli rientri nella spesa limite di 700 euro, perché è questa la miseria che con la vostra stravagante fantasia avete deciso di concedere a quei cittadini, proprio a loro che sono noti per la grande capacità di rimboccarsi le maniche e ripartire con grande forza, con più forza di prima. come definire il vergognoso botta e risposta del vice ministro Bignami con i sindaci del territorio? I titoli della stampa erano «Bignami minaccia gli alluvionati», è davvero pessimo leggere di un Vice Ministro incapace di accettare critiche rispetto al proprio operato e meno male che lui è uno dei migliori, almeno così vi sentiamo dire continuamente. Immaginiamoci gli altri come sono. Come risposta, poi, alle esigenze dell'area dei Campi Flegrei, avete deciso di trasformare un provvedimento *ad hoc* in un emendamento da inserire nel decreto-legge che stiamo votando oggi, un segnale molto chiaro - diciamocelo - dell'importanza che date a quella comunità e a quei territori. Come ricordato dal senatore Nave nell'intervento precedente, per dare un sostegno al tessuto economico in difficoltà abbiamo proposto diverse soluzioni, tra cui l'istituzione di una zona franca urbana, la decontribuzione Sud al 100 per cento invece che al 30 per cento, la cassa integrazione in deroga. di incrementare le risorse a disposizione, soprattutto per la messa in sicurezza delle scuole, e di prevedere dei fondi aggiuntivi per il consolidamento del nostro immenso patrimonio archeologico, ma a voi queste proposte non sono chiaramente piaciute. In Commissione, inoltre, avete respinto gran parte degli emendamenti delle opposizioni che assicuravano anche ai territori alluvionati dell'Emilia-Romagna e a quelli interessati dal fenomeno del bradisismo la possibilità di usufruire del superbonus rafforzato; emendamenti che avevamo predisposto per riparare al vostro errore del taglio della cessione del credito e dello sconto in fattura. Avete scelto, però, di farlo solo per il cratere dell'Aquila. Ci mancherebbe, per carità, da abruzzese ho apprezzato questa misura e personalmente l'ho sostenuta e votata; ci tengo a farvi notare che avete creato una incomprensibile disparità di trattamento tra i cittadini e i territori che vivono situazioni di difficoltà similari, seppur dovute a situazioni ed eventi diversi. diversi. In quasi due anni di Governo, non avete raggiunto alcun risultato utile, se non per il vostro ego e la vostra delirante narrazione. In Europa lottate per un commissario dicendo di mandarci Fitto, che con il PNRR ha fatto faville, salvo poi leggere quanto dice la Ragioneria generale dello Stato, che vi invita ad essere più cauti con i trionfalismi. Meloni fa festa ad ogni rata del PNRR che ci viene assegnata, dicendo che siamo arrivati al traguardo prima degli altri; non dice però quello che afferma la Ragioneria dello Stato,

Pensiamo al merito, che la signora Meloni poneva a base della sua e della vostra azione, anche per riscattare quanti, a suo dire, sono stati per decenni costretti ad abbassare la testa. Lo diceva poco prima delle elezioni,

chi doveva rialzare la testa: forse quei giovani di Fratelli d'Italia che volevano intascarsi i soldi del servizio civile, che abbiamo visto in quei vomitevoli filmati, o i Ministri indagati per truffa ai danni dello Stato? *(Applausi)*. Chi doveva rialzare la testa, il vice ministro Bignami che minaccia gli alluvionati,

forse prima di rialzare la testa, avrebbero dovuto riempirla, concedetemelo. *(Applausi)*. Qualcuno, quasi per giustificare e sminuire questi fatti, ha detto che queste cose aiutano la minoranza. No, cari miei, non ci siamo proprio: queste cose non aiutano noi. Queste cose qualificano voi e questa è cosa ben diversa. *(Applausi)*. L'unica azione concreta che avete che avete deciso di mettere in campo in questi mesi, tramite la Regione Lombardia, è stata l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Sapete bene come la pensa il Movimento 5 Stelle sulla questione, ma oggi vorrei fare un passo in avanti e venirvi incontro. Con l'aeroporto intitolato a Berlusconi avete di fatto liberato una nuova casella per l'intitolazione del Ponte sullo Stretto. Ed ecco il nostro suggerimento: intitolare il Ponte al noto Marcello Dell'Utri, come riconoscimento per aver fatto - lui sì il collegamento stabile con la Sicilia per anni e da ben prima che il progetto del Ponte si concretizzasse. *(Applausi)*. Magari assicurategli anche una rendita dei pedaggi, visto che per i prossimi anni dovrà dovrà accontentarsi solo della modesta cifra ricevuta grazie alla generosità di un anonimo donatore (chissà chi sarà). Lui se lo merita e se lo aspetta, lo capiranno, ne siamo certi. Anche nel provvedimento in esame sul merito vi siete superati. Penso all'articolo sulla Fondazione Milano Cortina che, grazie ad un'inchiesta, abbiamo scoperto essere rifugio per il riscatto lavorativo di giovani altamente meritevoli provenienti da famiglie in disagio economico. Ma non vi vergognate per niente di quello che state facendo? Ovviamente sono stata sarcastica con questa affermazione, ma non vi vergognate?

Presidente, io la ringrazio, per un minuto. Noi votiamo contro questo provvedimento, che riteniamo del tutto insufficiente. È esattamente come voi: è fatto di *slogan*, di parole distanti anni luce dai problemi del Paese reale; un Paese che state governando a vostra immagine e per quello che quotidianamente dimostrate di essere nella sostanza, nella forma e pure nel merito. È il peggior Governo degli ultimi decenni. *(Applausi. Commenti)*. Votiamo contro perché non siamo abituati a prendere in giro le persone, specie se sono in difficoltà.

Presidente, colleghi e Governo, ritorniamo a parlare del decreto-legge, perché il precedente intervento è stato solo un insulto continuo alla *Premier* e ai membri del Governo e nulla ha citato del provvedimento in esame. Il provvedimento oggi in votazione è invece la plastica dimostrazione dell'operatività e della fattività di questo Governo, che non si limita a fare promesse o provvedimenti *spot* - come siamo stati abituati in precedenza - limitati al momento dell'emergenza o finalizzati a colpire e impressionare positivamente l'opinione pubblica; ma quelle promesse le attua e le mantiene, dando continuità e costanza al suo lavoro. lavoro. Era il gennaio scorso quando intervenivamo con nuovi sostegni per i territori colpiti dalle alluvioni del maggio 2023, prevedendo, da un lato, aiuti per la ricostruzione e, dall'altro, aiuti per la ripartenza aiuti per la ripartenza delle industrie. Mentre a febbraio dell'anno prima approvavamo il decreto ricostruzione per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia e da quello dell'Aquila, con misure che semplificavano e acceleravano le procedure di ricostruzione. Adesso torniamo a occuparci di queste problematiche, con nuovi importantissimi interventi, che certamente potranno favorire la rinascita delle aree ferite innanzitutto dagli eventi alluvionali, aiutando la ricostruzione non solo degli edifici privati, ma anche di quelli pubblici, delle infrastrutture viarie e ferroviarie, delle opere di difesa idraulica e della rete dei servizi essenziali. Per farlo partiamo da una norma assolutamente innovativa, contenuta nell'articolo 1, cioè la previsione di contributi per i danni ai beni mobili distrutti o danneggiati dall'alluvione all'interno delle abitazioni private. Non era mai successo finora che un Governo si preoccupasse anche di questo, e cioè della mobilia, degli arredi, di tutto ciò che fa di una casa la nostra casa e che rappresenta qualcosa di essenziale per rendere quella casa abitabile e fruibile e la nostra vita una vita quotidiana, normale. Per la prima volta questa maggioranza pensa anche a questo aspetto, finora sempre trascurato, per quanto importantissimo, e dà la possibilità, a chi nell'alluvione ha perso tutto, di fruire di altri piccoli ma utilissimi sostegni. Questa previsione dimostra anche, più di ogni altra, quanto siano la sensibilità e l'attenzione che chi ha in questo momento nelle proprie mani le sorti dell'Italia mette nel guidarla, curando perfino dettagli che potrebbero essere insignificanti, ma che insignificanti non sono. Viene poi previsto che i contributi per la ricostruzione privata possano essere anche destinati alla delocalizzazione o all'acquisto di aree alternative o di immobili dove riavviare l'attività produttiva o fissare la nuova residenza, attraverso l'accelerazione delle procedure di ristoro, per garantire quanto prima il rientro nelle case di abitazione. In questo caso, le aree degli immobili demoliti, da demolire o comunque danneggiati, che vengono abbandonate da chi delocalizza la propria residenza, vengono acquisite gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune. Tutto questo avverrà sotto la stretta sorveglianza del commissario straordinario, con verifiche a campione, per le quali potrà avvalersi anche di enti pubblici o di organi statali con competenze ispettive di controllo e di vigilanza, per la prevenzione o la repressione di illeciti correlati all'utilizzo dei contributi pubblici. Anche questa norma è di fondamentale importanza, perché siamo stati normalmente siamo stati normalmente abituati a concedere soldi a pioggia ai territori che spesso non li utilizzano come dovrebbero o non li utilizzano appieno, perché sono mancati i controlli e le relative sanzioni. Con l'assegnazione di questo compito al commissario si può invece intervenire in maniera efficace anche sotto questo punto di vista e - perché no - agire anche culturalmente sulla mentalità e i comportamenti di chi magari pensa di poter profittare di finanziamenti pubblici per scopi diversi da quelli previsti, che sono la sono la restituzione della dignità a chi ha visto la propria normalità stravolta da una catastrofe naturale. La discussione del decreto-legge si è concentrata molto sugli aspetti finanziari. Siamo riusciti, con diversi emendamenti, a incrementare le risorse da destinare a territori e famiglie, mettendo particolare attenzione nella programmazione della spesa. Quindi diventa ancor più importante vigilare sull'impiego di queste risorse, ma anche accelerare la ricostruzione, il che si può fare solo attraverso una definizione più attenta delle relative modalità di attuazione. Ad esempio, si consente agli enti locali di poter assumere personale attraverso lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi o estendendo il novero dei soggetti che possono essere individuati quali soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. C'è poi tutto l'aspetto di intervento sulle infrastrutture ferroviarie e viarie, fondamentali per la ripresa di qualunque territorio. In questo caso, l'articolo 6 inserisce quelle ferroviarie nel piano speciale predisposto dal commissario straordinario e vengono previsti RFI, come soggetto attuatore per provvedere alla messa in sicurezza e ripristino degli impianti ferroviari ferroviari danneggiati, e l'ANAS, quale corrispondente soggetto attuatore per le arterie statali. Anche qui c'è un'attenzione mirata a voler far davvero ripartire le aree alluvionate attraverso l'affidamento di questi lavori a soggetti che sono garanzia per una buona riuscita degli interventi. Con questo provvedimento il Governo non ha trascurato le altre popolazioni vittime di calamità e catastrofi naturali o comunque a rischio. Per questo inserisce misure anche per l'area dei Campi Flegrei e per le zone terremotate. Per quanto riguarda i Campi Flegrei, anche in questo caso le nuove norme di protezione civile e prevenzione del rischio bradisismico si collocano nel solco della continuità con le previsioni già introdotte in precedenza, facendo un passo in avanti quanto a utilità e importanza. Tra le varie previsioni, viene introdotta la nomina di un commissario straordinario, in carica fino al dicembre 2027, per assicurare la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica e la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. Vengono poi introdotte una serie di misure di semplificazione, accelerazione e deroga alle procedure esistenti per l'attuazione degli interventi, nonché misure emergenziali per assicurare la continuità scolastica, per esempio dei bambini e i ragazzi della zona, così che non siano penalizzati nel loro percorso di studi. Inoltre, si torna a pensare anche alle popolazioni colpite dal terremoto dell'Aquila nel 2009 e del Centro Italia del 2016, con misure che potenziano alcune aree di intervento. Alcune di tali misure sono un ulteriore mattoncino - per usare un termine che cade a pennello visto l'argomento - nella ricostruzione di quelle aree e dimostrano, se ce ne fosse bisogno, l'efficacia di questo provvedimento. Voglio cogliere l'occasione per sottolineare anche alcuni aspetti, come ad esempio gli ottimi risultati raggiunti in questo ambito sotto la nostra legislatura. Nonostante i problemi sopraggiunti che rallentano l'attività di ricostruzione come lo stesso commissario ha recentemente ricordato, e mi riferisco all'inflazione, all'aumento dei costi dei materiali, alle difficoltà di approvvigionamento, alle difficoltà di trovare le maestranze e così via - questo Governo è riuscito, con un suo intervento, a dare una spinta decisiva alla ricostruzione stessa. I dati che voglio citare, che sono dell'ultimo rapporto dell'ufficio commissariale - parliamo di numeri, giusto per rispondere

che ci dice che, al 30 giugno, sono stati concessi quattro miliardi e mezzo di euro, di cui, nel solo 2023, è stato erogato un terzo del totale e, nell'ultimo biennio, addirittura il 50 per cento dell'intero ammontare, quindi con un continuo *trend* in crescita segnato nei primi mesi dell'anno. il cambio di passo rispetto al passato. Si è finalmente innescato un percorso virtuoso. Per citare sempre il rapporto, gli ultimi dati illustrano una forte fluidificazione del sistema di ricostruzione dopo molti ritardi accumulati negli anni nel post sisma. La nomina dei commissari, signor Presidente - per rispondere alla senatrice Furlan - non può essere associata alla bontà o meno del codice degli appalti, perché nulla c'entra, ma a volte serve. Qui stiamo parlando di programmi straordinari di ricostruzione. Serve a garantire una risposta più efficiente e più tempestiva nelle operazioni di ricostruzione. Quindi, credo che, alla luce di tutto questo, nessuno potrà mai smentire l'eccezionale lavoro che questo Governo sta portando avanti in tema di calamità naturali: che siano alluvioni, che sia il sisma, che sia la prevenzione del rischio, riuscendo

del tempo. Stiamo intervenendo concretamente, con i provvedimenti già varati e con questo decreto e gli altri che arriveranno. Per tutte queste ragioni, esprimo il voto favorevole del Gruppo Lega a questo provvedimento.

Questo è stato l'evento alluvionale in Emilia-Romagna di più di un anno fa. Basterebbero solo questi numeri a richiederci sufficiente serietà, responsabilità e i giusti toni, e cioè di muoverci nel segno della collaborazione e della determinazione comune negli interventi, anche per rendere ai cittadini la percezione di un solo Stato al loro fianco, non di mille articolazioni che litigano tra di loro. è anche il miglior modo di rendere onore alla resilienza e alla laboriosità di un popolo che si è rialzato da solo, al fianco delle proprie amministratrici, dei propri amministratori locali, delle Forze dell'ordine, delle associazioni dei volontari. signor Presidente, siamo costretti a non tacere il cinismo di un Governo che, dal primo giorno ad oggi, ha immaginato di utilizzare questo evento come la possibilità di un assalto alla diligenza, come una possibile strumentalizzazione elettorale. *(Applausi)*. Bisogna dire la verità: gli stivali nel fango del presidente Meloni, la promessa del 100 per cento la polemica quotidiana a tutto campo con gli enti locali avevano questo obiettivo. Ripeto: diciassette morti e 20.000 sfollati, all'inizio erano 36.000, miliardi di danni stimati, il terzo evento calamitoso più grave nel mondo nel 2023. Oggi, d'altra parte, c'è stata una dimostrazione plastica. Mi ha molto sorpreso la relatrice, che in Commissione ha avuto toni di confronto, che oggi invece ha fatto sostanzialmente un comizio elettorale, in particolare contro il sindaco di Ravenna. Signor Presidente, faccio una premessa. Io vorrei davvero sorvolare sulla confusione totale che, come ha detto il senatore Manca, abbiamo tristemente osservato in queste settimane: non solo l'incontinenza in materia di decretazione d'urgenza, facendo ancora una volta finta che il Capo dello Stato non abbia parlato in merito, ma il capolavoro al contrario. Noi convertiamo, infatti, due diversi decreti confluiti, uno dei quali, quello sui Campi Flegrei, su una materia già oggetto di decretazione di urgenza pochi mesi fa e che oggi, con questo provvedimento, è completamente sostituito. Poi, cito i pareri arrivati in ritardo, subemendamenti a ripetizione e infine infine pareri sostanzialmente tautologici nella Commissione. A fronte dei nostri emendamenti e delle nostre proposte, la risposta è: o che non fa parte del programma del Governo, oppure che il MEF indica che per alcuni emendamenti c'è una copertura, mentre per altri no. In questo caso è del tutto evidente che nel secondo caso è una scelta. È qui lo sforzo che sia la relatrice sia la Sottosegretaria hanno fatto, con un Governo poco collaborativo. Insomma, è la dimostrazione che il Parlamento è stato sostanzialmente esautorato. Poi, nel merito, noi abbiamo avuto sempre un'unica stella polare, quello che avete detto voi alle popolazioni di quei territori: avrete il 100 per cento dei ristori. La risposta che oggi c'è è positiva? No, è negativa. Non li avranno: questo è il punto. *(Applausi)*. Vorrei dire un solo numero:

Voi avete detto che i Comuni non hanno speso ancora tutte le risorse, ma ai Comuni abbiamo dato le risorse per ricostruire strade e ponti; devono attenersi al codice che prevede procedure e che pure i Comuni hanno rispettato in tempi record e che adesso stanno appaltando. si è istituita una cabina di regia tra Stato ed enti locali, ma non l'avete mai riunita. Io ho fatto un'esperienza nella mia vita, quando ero molto giovane: terremoto dell'Aquila del 2009, presidente del Consiglio Berlusconi, sottosegretario Bertolaso. Noi ci riunivamo la mattina alle ore 7, la sera alle ore 23, dal primo giorno e per mesi tutti tutti i giorni, enti locali, Forze dell'ordine, Forze armate, grandi società nazionali per l'energia e per il gas; abbiamo gestito insieme quell'evento, pur da parti politiche completamente distanti. distanti. Quella cabina che non avete mai riunito è il luogo in cui chiarirsi con gli enti locali, evitando la polemica, o almeno che la polemica non sia il fine. Allora, il tema del rapporto Governo-Comuni qui merita un approfondimento, perché la senatrice Valente ha ricordato che il ministro Musumeci, proprio ieri sui Campi Flegrei, ha detto che tutta la responsabilità è dei Comuni. Qui abbiamo sentito che tutta la responsabilità è dei Comuni. Ora il dubbio sorge spontaneo: esattamente qual è la vostra idea di autonomia differenziata? A me pare che l'unica differenza sia questa: quando si tratta del provvedimento "spacca Italia" - naturalmente so che quando dico questo i colleghi della Lega non si scompongono, anzi ne menano vanto, mentre quelli di Fratelli d'Italia masticano amaro

e migliaia di banchetti, promossi da partiti, sindacati e associazioni, stanno riempiendo le nostre piazze: un enorme «no» vi travolgerà. Questa è l'autonomia differenziata "spacca Italia". Quando invece si tratta dei Comuni, cioè dell'autonomia locale più antica e riconosciuta dell'Italia, voi ne fate bersaglio per le vostre Noi siamo completamente contrari all'idea che ci sia un vittimismo di Stato che scarichi sempre la colpa a qualcuno, che ci sia uno scaricabarile verso le autonomie locali soprattutto, siamo contrari proprio all'idea che ci possa essere un Sottosegretario che vada nei territori colpiti e dica, per coloro che sono eterodiretti dal PD, che non si sa se ci saranno i 6.000 euro che nemmeno bastano a proposito di come si affronta un evento così drammatico. Avete trattato le amministrazioni locali come dei questuanti, quando invece il Paese dovrebbe dotarsi della certezza del diritto, di quel codice della ricostruzione adesso in discussione alla Camera. Lo aspettiamo in Senato, ma lo aspettavamo da due anni. Io vorrei dire che c'è un tema tutto politico. È un suggerimento non richiesto: si può, dopo aver vinto le elezioni, dire che è colpa dei Governi precedenti e che si sta facendo di più dei Governi precedenti? Tuttavia, è una formula che scade come lo yogurt. non a noi dovete rendere conto, ma a quelli che vi hanno votato, ai quali, se continuate a dire che il problema sono i Governi precedenti, a un certo punto vi chiederanno che vi hanno eletto a fare: a governare il Paese o a continuare a fare opposizione a quelli che c'erano prima? Certo che ci sono fenomeni enormi come il caos climatico, che moltiplicano gli eventi climatici estremi. Tutte le volte che ne abbiamo discusso e abbiamo parlato di transizione energetica ci avete raccontato che il problema era la Cina. Penso che la presidente Meloni sia andata in Cina a dire questo, che il problema sono loro. Ieri la senatrice Petrucci si è lanciata, con sprezzo del pericolo, nell'indicazione della soluzione a tutti i problemi: il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima che avete approvato, il PNIEC. di quel pezzo di carta nel quale avete scritto che tutti i nostri problemi saranno risolti dal nucleare: la nuova generazione della fissione nel 2035, forse, e poi la fusione nel 2050, quindi coloro che osservano e rispondono ai fenomeni climatici estremi oggi aspettino con calma che arrivi Poi, a proposito del dissesto, la senatrice Petrucci ha detto che il Governo ha scritto a tutte le Regioni e solo sei hanno risposto. Ora, io per gentilezza non dirò quali sono le sei Regioni che hanno risposto. Certamente non penso che il Governo abbia una

La verità è che la calamità non è l'oggetto di questo provvedimento: è il soggetto. Siete voi la calamità. Questo è il punto! *(Applausi)*.

poco si vota in Emilia-Romagna e anche in altre Regioni. Si vota in quei territori colpiti, e voi avete attaccato oggi qui Michele De Pascale, che invece ha detto una cosa giusta: tra gli interventi manca completamente la voce della prevenzione e della messa in sicurezza. Purtroppo l'evento che si è verificato non va guardato con gli occhi del passato, ma con quelli del futuro. È un evento straordinario per il passato ma nessuno, visti i cambiamenti climatici, ha il coraggio di parlare abbastanza di straordinarietà guardando al futuro. Bene vedremo vedremo infine, proprio in quel momento, dopo che avete vantato tante volte il voto alle politiche, a chi daranno ragione le cittadine e i cittadini di cui voi non vi siete occupati a sufficienza e che alla fine vi giudicheranno.

Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ritengo inaccettabile ascoltare nell'Aula del Senato un intervento come quello della senatrice Di Girolamo, privo di qualsiasi contenuto utile alla discussione, pieno esclusivamente di inaccettabili offese. Evidentemente qualcuno ha scambiato la Camera alta per un *cabaret*. il senso delle istituzioni non appartiene a tutti noi. Voglio nuovamente ribadire la vicinanza del Gruppo Fratelli d'Italia a tutte le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana, delle Marche e dei Campi Flegrei, che stanno affrontando una difficile situazione. E desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e a tutte le donne che stanno lavorando per il ritorno alla normalità. Ringrazio i volontari, la Protezione civile, gli amministratori locali, i sindaci *(Applausi)*, le Forze dell'ordine e il commissario alla ricostruzione, il generale Figliuolo. Speravo che questa discussione potesse essere serena e concreta e non influenzata dall'imminente campagna elettorale in Emilia-Romagna, ma evidentemente così non è stato. Ho sentito dire durante il dibattito che questo provvedimento sarebbe assolutamente privo di copertura economica, che in questo primo anno non si è visto nulla e che le risorse stanziate non sono sufficienti. E allora mi preme ribadire che il Governo da subito ha dato prova di tempestività, esprimendo la chiara volontà, che ribadiamo quest'oggi in Aula, di dare ristoro al 100 per cento dei danni subiti dai privati. Ad oggi il Governo ha stanziato, di concerto con la struttura commissariale, 4,7 miliardi per la ricostruzione, di cui 2,8 miliardi per le opere pubbliche e 1,9 miliardi per la ricostruzione privata.

sono serviti per un bilancio del primo anno del commissario Figliuolo. Ho letto in una sua dichiarazione comparsa sui giornali che dai dati raccolti finora si può affermare che tali risorse permettono di far fronte a qualsiasi esigenza. *(Applausi)*. Nonostante tutto, il centrosinistra continua a raccontare una verità che non trova riscontro nella realtà. Abbiamo anche assistito a un gioco al rialzo, che è continuato anche questa mattina in Aula. Come sapete, il decreto in esame destina a una platea di 35.000 soggetti un contributo massimo di 6.000 euro ad abitazione per risarcimento dei mobili distrutti dall'alluvione. In Commissione - come dicevo quest'oggi in Aula sull'argomento durante la discussione degli emendamenti, abbiamo assistito nuovamente a una sorta di gioco al rilancio. Dalle opposizioni con gli emendamenti c'è chi proponeva 12.000 euro, chi 18.000, chi 30.000. Peccato, che quando si è trattato del sisma del 2012 dell'Emilia-Romagna, i Governi di centrosinistra, il commissario Bonaccini, non hanno stanziato nulla per i beni mobili. *(Applausi)*. Nulla per i beni mobili! Certo, il centro sinistra e, in special modo, il MoVimento 5 Stelle se ne intendono di arredamento, considerando che hanno speso 100 milioni di euro per i banchi a rotelle. Ad un anno dalla nomina del commissario Figliuolo per le opere pubbliche sono stati realizzati oltre 6.000 interventi sulla viabilità, sul reticolo idrico, su argini e fiumi. Il 35 per cento degli interventi è stato ultimato, il 30 per cento è in fase di progettazione e così si andrà avanti fino a coprire il 100 per cento dei lavori pubblici. Nelle settimane successive all'alluvione sono stati erogati i contributi di immediato soccorso. Come ricordava prima il collega Lisei, 23.000 famiglie hanno ricevuto in media 5.000 euro, con uno stanziamento di 103 milioni di euro. Anche questa è una novità mai vista in passato. Certo, bisogna continuare a lavorare per fare ancora meglio, incentivando in particolare i privati nella ricostruzione, ma certamente le accuse di aver fatto passerelle o di aver mentito alle popolazioni le rispediamo sonoramente al mittente. Il Governo Meloni ha dato prova di grande concretezza e tempestività rispetto alle emergenze e con i decreti in esame intendiamo ulteriormente velocizzare i processi di ricostruzione, estendendo la platea dei soggetti attuatori degli interventi di riparazione. data la possibilità agli enti locali di potenziare l'organico amministrativo. Abbiamo introdotto con un emendamento di Fratelli d'Italia una norma fondamentale che agevola la ricostruzione del sisma 2009. I Campi Flegrei rappresentano un'altra emergenza per l'Italia, dove convivono contemporaneamente - come ha ricordato recentemente il ministro Musumeci ministro Musumeci - i rischi sismico, vulcanico e il bradisismo. È opportuno ricordare che in pochi mesi è la seconda volta che torniamo ad occuparci di questo argomento in Aula proprio a dimostrazione dell'attenzione che il Governo Meloni e il ministro Musumeci hanno nei confronti dei cittadini dei Campi Flegrei. Negli ultimi anni si è fatto molto di più rispetto agli ultimi ottant'anni. Oggi, dopo il forte evento sismico del 20 maggio, si propongono ulteriori interventi, ma è un'area che purtroppo paga anni di gravi irresponsabilità nella gestione del territorio. In questa zona si è continuato a costruire come se il bradisismo non esistesse. Trovo assurdo che, nonostante le evidenti pericolosità ambientali, nessuno si sia fatto mai di limitare l'aumento del carico urbanistico. Lo abbiamo fatto noi con questo decreto-legge, vietando il rilascio di titoli edilizi per interventi di nuova costruzione. *(Applausi)*. Questa è la verità che fa male alle opposizioni. Il decreto prevede la nomina di un commissario straordinario al fine di attuare interventi di riqualificazione sismica sugli edifici pubblici e garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e dei servizi fondamentali; si prevedono procedure semplificate per la progettazione e per la realizzazione degli interventi come quelli di ripristino e di riqualificazione sismica degli edifici. Viene autorizzato un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Viene stabilita la procedura per l'adozione di un piano per la riqualificazione sismica del patrimonio privato con contributi per la riparazione degli edifici privati. oggi ho sentito parlare del tema della delocalizzazione degli edifici situati in zona di alta pericolosità. Più volte ho sentito, sempre oggi, parlare della necessità in queste aree di provvedere all'adeguamento sismico del patrimonio immobiliare. Le opposizioni solo oggi si sono accorte di queste problematiche. Chiedo per suo tramite, Presidente, ancora una volta all'opposizione perché non ha affrontato questi temi quando erano al Governo. Perché non avete finalizzato il vostro superbonus al miglioramento sismico o alla delocalizzazione degli immobili in queste aree ad alta pericolosità? Avete speso 220 miliardi creando un buco alle casse dello Stato, altro che lettere! Solo cambiali ci avete lasciato per un grande *spot* elettorale, consentendo di ristrutturare gratuitamente ville e castelli in ogni parte d'Italia senza occuparvi dei veri problemi della Nazione. Il superbonus è stata un'autentica follia, di cui portate la responsabilità politica ed oggi vi permettete di salire sul pulpito per elargire insegnamenti su come mettere in sicurezza il territorio nazionale. Non siete credibili. Il Governo Meloni e il ministro Musumeci continueranno a lavorare per mantenere gli impegni presi, dando risposte certe alle popolazioni colpite dall'alluvione e dai sismi e ai residenti dei Campi Flegrei. Signor Presidente, con questo mio intervento annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

senatore Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Stiamo però parlando della senatrice Zedda.

che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici ed è composto di due articoli. L'articolo 1 reca disposizioni volte a prorogare il termine di adozione dei testi unici

questa Presidenza non lo tollererebbe.

uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione dei testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, ovvero non più attuali. La disposizione in esame proroga il termine di adozione dei sopracitati testi unici dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025. Nell'analisi dell'impatto della regolamentazione si evidenzia che sono ancora in corso di lavorazione i decreti delega in materia di IVA e tributi degli enti territoriali. Peraltro, devono ancora essere definitivamente approvati i decreti delegati recanti disposizioni nelle seguenti materie: riordino del sistema nazionale della riscossione; revisione del regime impositivo dei redditi, dell'imposta di bollo e di altri tributi indiretti diversi dall'IVA; revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, che dirvi? Il Governo chiede di avere una delega per il riordino dei testi unici in materia di tributi e si dà un termine da solo: chiede di avere tempo fino al 29 agosto 2024. Dopodiché, si rende conto di non arrivarci e allora presenta un'altra legge e dice "datemi un ulteriore termine, anzi mi prendo un ulteriore termine e mi impegno a portare a casa questo risultato, nei modi in cui riuscirò a farlo, entro il 31 dicembre 2025". Se consideriamo che la legge delega era stata fatta nell'agosto 2023, stiamo parlando di un bel tempo in avanti, oltre due anni e mezzo di tempo per il riordino dei testi unici.

di anno in anno si susseguono e vengono varate e approvate dal Parlamento *ad hoc* su determinati provvedimenti. Sono certamente testi disorganici, composti da provvedimenti che si susseguono negli anni.

non può non attirare da parte delle opposizioni almeno un giudizio critico e un richiamo a una maggiore attenzione e a un maggiore rigore, per due motivi. Il primo

forse, in senso ancora più pratico, questa continua produzione di decreti-legge che si susseguono uno dietro l'altro, anche quando non ci sarebbe motivo di ricorrere alla decretazione d'urgenza,

ormai in contrasto con la legislazione dell'Unione europea, dunque con norme sovraordinate che le pongono fuori dall'ordinamento), non riesce a rispettare il termine. Questo dovrebbe essere un motivo per il Governo, ma anche per le forze dell'opposizione, per fare una seria riflessione su questi primi due anni di Governo e di legislatura e per rendersi conto che quello che diciamo come forze dell'opposizione quando critichiamo il ricorso continuo alla decretazione d'urgenza non ha semplicemente una ragione politica e non è una mera critica politica, ma è anche una critica a questo che non consente di avere una produzione legislativa ordinaria e soprattutto ordinata, perché pecca di mancanza di sistematicità e di organicità. Quando in un testo come quello che abbiamo appena votato sulla protezione civile ci troviamo le norme anche sui grandi eventi sportivi, sulle Olimpiadi di Milano Cortina, insieme alle norme sui Campi Flegrei, insieme alle norme sulle alluvioni e sui rimborsi per l'acquisto dei beni mobili, è chiaro che sulla *Gazzetta Ufficiale*

Se non basta un anno e mezzo e ci vuole un ulteriore anno e mezzo per fare semplicemente un'opera di pulizia di testi unici già esistenti, significa che è arrivato il momento che il Governo si renda conto che continuare a fare decretazione d'urgenza porterà semplicemente a un affastellamento di norme di vari argomenti, a una produzione eterogenea che non ha un'organicità e che non può essere né eseguita, né applicata correttamente. Questo vale a maggior ragione per quanto riguarda il regime dei tributi: ricordo che già con la scorsa legge di bilancio è stato introdotto il taglio del cuneo fiscale, ma come misura temporanea. Il ministro Giorgetti ci ha annunciato che verrà applicato anche per la prossima legge di bilancio, quindi vi saranno due esercizi finanziari con una misura che non c'era prima e che non sappiamo se verrà applicata stabilmente (al momento è una misura temporanea).

la compilazione del suo modello di dichiarazione dei redditi, saprà che fino a un certo anno c'era un regime tributario, dal 2023 in poi ce n'è stato un altro e forse proseguirà per il 2024 (anche perché ricordo che il nostro sistema

o quantomeno un'incertezza interpretativa, anche nella misura in cui dovranno essere fatti poi gli accertamenti e le verifiche sulle dichiarazioni dei redditi. Anche l'Agenzia delle entrate si trova quindi davanti a disposizioni di durata temporanea, il che significa che, nel ricostruire la posizione di un contribuente, saprà che fino a un certo periodo dovrà applicare un determinato regime e per gli anni successivi ne dovrà applicare altri. Voi capite che questo sistema e questo modo di lavorare, anche dal punto di vista della legislazione in tema tributario e fiscale, intanto generano confusione nel contribuente, incertezza applicativa per l'operatore che lo deve assistere

facilmente interpretabile o, quantomeno, facilmente consultabile. L'Agenzia delle entrate, in adempimento alle disposizioni di questa legge delega, ha reso consultabili sul suo sito,

i nuovi testi disponibili, perché nel frattempo il Governo ha continuato a modificare la normativa. Penso anche, signor Presidente, alle varie rottamazioni che ha fatto questo Governo; che pure vanno a incidere. Anche sulla riscossione c'è una proposta

tributaria, che è uno strumento a sé, e con le nuove norme sulla dichiarazione dei redditi. In tutto questo, il Governo continua a fare decretazione d'urgenza e e cambierà le norme anche per il prossimo anno. In legge di bilancio, infatti, è stato anticipato che verrà rinnovato il cuneo fiscale come misura temporanea. Nel frattempo, però, questi testi unici sono ancora in attesa. Forse, entro dicembre 2025 verranno finalmente pubblicati o, più probabilmente, quando verranno pubblicati già saranno oggetto di emendamenti, perché il Governo, nel frattempo, avrà fatto altri decreti-legge, altre leggi temporanee o altre misure non dotate di lungimiranza e di programmazione, che renderanno vano anche questo lavoro.

durante la discussione sulla cosiddetta riforma tributaria, abbiamo votato contro, perché dicevamo che l'impostazione era sbagliata e pasticciata. Il Governo,

mezzo. La domanda allora è cosa si è fatto: a che punto siamo? Per quale ragione bisogna fare la proroga? Bisognerebbe dirlo. Quali intoppi si sono trovati?

Addirittura, si vuole fare la *flat tax*. Penso invece che si dovrebbe affrontare il tema che chi più ha più deve pagare, con una grande scala e gradini e gradini anche molto vicini tra di loro, per fare in modo che ognuno paghi il giusto. Perché serve avere un sistema tributario che funzioni?

quando avete deciso di accelerare, l'avete fatto con decreti-legge. Lo avete fatto in precedenza e probabilmente lo farete anche domani: siamo chiamati a tempi stretti e a fiducie una dietro l'altra, che impediscono la discussione. Forse è giunto il momento

chi più aveva continua ad avere di più e chi meno aveva continua ad avere di meno; sostanzialmente, il sistema tributario fa acqua da tutte le parti. Intervenire è quindi necessario e urgente,

perché in questi primi interventi dei colleghi si contesta oggi una cosa che non è mai esistita e non è mai stata fatta nella storia repubblicana di questo Paese: dopo cinquant'anni, una seria riforma del fisco, una seria riforma fiscale; mai nessuno ci aveva messo mano. Questo Governo, in un anno e mezzo, ha fatto passi da gigante *(Applausi)* e, nonostante questo,

i testi unici che la riforma fiscale chiede: ne sono già stati approvati tre e sono appunto quello sulle sanzioni tributarie, amministrative e penali, quello sui tributi erariali minori e il testo unico sulla giustizia tributaria. Quindi serve un po' di tempo, perché bisogna fare la ricognizione oggi di migliaia e migliaia di norme che oramai, nel sistema fiscale, si sono stratificate in tutti questi anni. Non è un'operazione semplice, da un punto di vista legislativo e normativo. Quella che il Governo sta affrontando è stata una priorità non soltanto del programma

tutti i contribuenti e non, come qualcuno in quest'Aula poc'anzi sosteneva, solo per alcuni. Sarà un vantaggio per tutto il sistema: lavoratori (autonomi, dipendenti o indipendenti) e imprese.

I testi unici che ancora mancano sono quelli relativi a imposte sui redditi, IVA, imposta di registro e altri tributi indiretti, agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori, adempimenti, accertamenti, versamenti e riscossioni. È importante

altro aspetto è relativo al fatto che oggi, in un anno e mezzo di Governo e in questa battaglia sulla riforma fiscale, sono stati già emanati 11 decreti fiscali per attuare la riforma del fisco attraverso quello che oggi dev'essere un rapporto di collaborazione tra il contribuente e il fisco,

La proroga, quindi, è necessaria per un riordino organico. Ecco perché serve il rinvio, proprio per assicurare l'organicità di tutta la materia e la completezza del quadro normativo.

tra Stato e cittadino. Le osservazioni che stanno arrivando sono numerose, molto dettagliate e puntuali, quindi si sta facendo anche questo tipo di lavoro di collaborazione. anche un'altra questione importante che è stata al centro del dibattito politico proprio in queste settimane: quello strumento vetusto, vecchio e impositivo, che entrava nelle case di tutti i cittadini che è stato il redditometro, grazie alla nostra battaglia, oggi finalmente è stato abolito. Basta con questo fisco opprimente. Forza Italia ritiene da sempre superata la logica del redditometro, quindi propone modelli come quello del concordato preventivo.

perché abbiamo chiesto con forza l'abolizione del redditometro, che era uno strumento vessatorio per il contribuente. Del resto, il recupero dell'evasione *record* che abbiamo avuto in questi anni - quasi 25 miliardi conseguenza di due anni di politica economica che ha posto le basi per una crescita sostenuta, accompagnata da un solido aumento dei posti di lavoro, che ha già fatto registrare il *record* di occupazione e il tasso più basso di disoccupazione degli ultimi quindici anni. Un gettito fiscale spontaneo dei contribuenti in misura così importante costituisce oggi una base solida su cui mettere le fondamenta della prossima legge di bilancio. Questi sono gli auspici, oggi, di una riforma fiscale che è iniziata che è iniziata e non si è mai fermata. Voglio ricordare che 11 decreti attuativi sono già stati emanati, tre testi unici già presentati ed altri comunque già pubblicati. Ecco perché non si sta perdendo tempo, anzi, si sta andando avanti in maniera spedita. La legge di bilancio, come dicevo, vedrà confermata la riduzione del contributivo sui redditi medio-bassi degli italiani, altre importanti misure di carattere sociale e un approccio più misurato e ragionevole al *deficit*, al contenimento del debito pubblico e alla programmazione del 2025 e degli anni successivi. Evidenziate

una vera e propria rappresentazione teatrale tragico-comica. Sarebbe stato forse meglio non mettere mano alla riforma.

cui si prevedeva di approvare i testi unici entro agosto 2024. Più volte il Governo e lo stesso Vice Ministro avevano annunciato addirittura l'approvazione prima dell'estate di ben dieci testi unici. Oggi apprendiamo che siamo all'anno zero. Vi accorgete anche del pasticcio, che noi avevamo evidenziato. Come si può procedere ad approvare dei testi unici con una riforma fiscale in corso di attuazione? *(Applausi)*. Questa era l'assurdità, che dimostra però la superficialità, l'approssimazione e la mancanza di programmazione, nel momento in cui vi accingete a realizzare delle riforme. È come se volessimo costruire un palazzo senza aver completato la progettazione esecutiva. È ciò che volevate realizzare con questo provvedimento. Oggi quindi ci chiedete questa ulteriore proroga. Attenzione, sono tanti i provvedimenti in cui dimostrate approssimazione e superficialità. Partiamo dal calendario fiscale: più volte lo avete modificato, promettendo, anche qui, la semplificazione. Oggi però i professionisti e i contribuenti si accorgono che siamo nuovamente nella congestione delle scadenze e dei pagamenti. Vi accingete

Prima è stato approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, poi la presidente Meloni lo ha sospeso e, in ultimo, lo state per reintrodurre

Questo significa concedere e riconoscere una vera e propria franchigia di evasione fiscale. *(Applausi)*. Non è così che si combatte l'evasione fiscale,

ridurre l'utilizzo del contante e soprattutto di andare a scovare le false residenze nei paradisi fiscali. Altro aspetto controverso di questa riforma il concordato preventivo biennale. Doveva essere il fiore all'occhiello di questa maggioranza e di questa riforma. Oggi, però, si sta trasformando in un fiore

Tremonti. Qui avete rispolverato dai vostri cassetti vecchi e impolverati una misura che già nasce fallimentare. Noi la contestiamo sul piano metodologico, perché non potete chiedere soldi a chi le tasse già le paga, ovvero i contribuenti affidabili, che hanno già un'affidabilità accertata, in base agli indicatori sintetici Nei confronti di questi contribuenti state introducendo l'istituto del ricatto, perché o accettano la proposta oppure subiranno verifiche.

Nei confronti di questi falsi contribuenti, di questi falsi cittadini, state promettendo tanti regali. Siete partiti riservando la possibilità di accesso prima ai contribuenti affidabili, poi vi siete accorti che questa misura non attirava le attenzioni dei contribuenti evasori, quindi l'avete estesa ai forfettari, concedendo loro addirittura un beneficio e un ulteriore regime agevolativo con una tassazione al 15 per cento, che per le *startup* si riduce al 3 per cento; inoltre, per rendere più appetibile la misura, avete concesso anche uno sconto del 50

poi il tema della pressione fiscale, altro obiettivo. Nel recente rapporto dell'Unione europea, il nostro è tra i primi Paesi con la pressione fiscale ancora più alta, pari al 42,7 per La pressione fiscale aumenta grazie all'aumento delle entrate tributarie che voi state vantando come risultato: +12 miliardi nel 2023 in base al rendiconto che è in corso di approvazione nell'assestamento prevedete +25 miliardi. Attenzione, però: a pagare queste entrate tributarie sono i soliti contribuenti (lavoratori, pensionati, imprese e lavoratori affidabili), perché gli evasori non concorrono a questo aumento delle entrate tributarie. Siete anche rimasti lontani dalle nostre proposte di far pagare un contributo di solidarietà a chi oggi sta realizzando extraprofitti, perché quelle entrate tributarie non derivano dalla tassazione degli extraprofitti. Nell'ultimo bollettino Consob di questi giorni, addirittura le banche quotate stanno realizzando extraprofitti per un +67 per cento rispetto all'anno scorso, passando da 15,7 a 26,2 miliardi. Rinnoviamo l'invito al Governo ad introdurre quanto prima una tassazione equa e giusta sugli extraprofitti non solo delle banche, ma anche delle assicurazioni e soprattutto delle imprese del settore delle armi, che stanno facendo

tra fisco e contribuenti: avete cancellato un istituto che permetteva, soprattutto ai piccoli contribuenti che incorrevano in qualche controversia con il fisco fino a 50.000 euro, di ricorrere alla mediazione, cioè a un terzo mediatore che cercava di fare sintesi. Ora avete escluso questi contribuenti da questo istituto. Il risultato è che nel primo trimestre del 2024 i contenziosi tributari sono aumentati del 38 per cento. Questo è uno dei fallimenti della vostra riforma. Vi ricordo che uno degli obiettivi del PNRR era ridurre il contenzioso tributario. Concludo, signor Presidente, dicendo che tutto ciò che è stato indicato e annoverato in questo mio breve intervento, dimostra il pressappochismo del Governo e a questo punto termino il mio intervento con la citazione di un noto critico teatrale statunitense, dato che stiamo assistendo a un vero e proprio teatrino fiscale. a George Jean Nathan, quando diceva che i cattivi rappresentanti sono eletti dai bravi cittadini che non votano. Esprimo pertanto la nostra contrarietà al provvedimento in

ampia e non settoriale, riguarda l'intero sistema fiscale e come tale è anche complessa, pertanto è giusto che le cose si facciano bene. È noto che l'ottimo è nemico del bene, quindi le cose vanno fatte con attenzione. In materia fiscale una virgola, un aggettivo, un termine cambiano la sostanza di una norma, quindi bisogna procedere con la giusta velocità, attenzione e fermezza ed è quello che esattamente stiamo facendo, tant'è che esprimeremo un ulteriore parere entro la chiusura estiva, poi riprenderemo a settembre con

una sessione, un mese, tre mesi l'anno, proprio a compilare testi unici. Questa sarebbe un'enorme opera di semplificazione che valorizzerebbe anche molto il lavoro delle nostre Commissioni. Ribadisco pertanto il voto favorevole della Lega al provvedimento

un po' ci obbliga - lo dico, per suo tramite, al presidente Garavaglia - a tracciare un bilancio della delega fiscale dopo un anno dalla sua approvazione in quest'Aula (erano i primi di agosto, i colleghi ricorderanno) e una decina abbondante di decreti legislativi dopo l'approvazione della delega. Quell'approvazione in quel momento, lo scorso anno, fu celebrata dal Governo Meloni come una rivoluzione in campo fiscale; una rivoluzione - oggi apprendiamo - che chiede la proroga, quindi è una rivoluzione meditabonda, che cammina a passo lento. Quella delega noi l'abbiamo contrastata lo scorso anno e durante il suo *iter*, per tre fondamentali ragioni, per tre fondamentali *vulnus* di impostazione e di principio che contiene. Il primo è il fatto che tutti i provvedimenti attuativi della delega sono una palese violazione del principio costituzionale di equità orizzontale, perché le misure dei decreti legislativi sono frammentarie, che parlano di regimi separati e di cedolari secche, non rispettando un principio di equità orizzontale che dovrebbe Il secondo grande problema è quello relativo al contrasto all'evasione fiscale. I decreti legislativi che abbiamo esaminato in Commissione parlano tutti una lingua ammiccante nei confronti di chi sceglie di evadere le tasse e di avere un rapporto di infedeltà fiscale. Questo è un altro grande tema che ci ha portato

tema, quello della tenuta dei conti pubblici. Tutte queste misure mettono gravemente in discussione e a rischio gli equilibri economico-contabili; è probabilmente questa la ragione del ritardo di cui oggi parliamo. Ci sono aspetti della delega - penso al riordino dell'IVA oppure alla revisione dei tributi degli enti locali - che non hanno ancora cominciato l'*iter* e non sono ancora stati visti dalle Commissioni del Parlamento (Camera e Senato), perché sono misure che hanno dei costi che evidentemente il Governo e il nostro Stato non possono permettersi.

che già soffriva di un grande e grave dualismo tra i contribuenti che sono assoggettati al pagamento dell'Irpef, che per definizione non possono evadere le tasse, e tutti quelli che hanno la possibilità, per la natura dei redditi che introitano, di essere assoggettati a regimi cedolari separati o a *flat tax*. Non si può tacere, a questo proposito, il richiamo che è già stato fatto dal collega Turco sui continui inciampi e sul fallimento cui è incorsa la misura simbolo di questa delega, delega, il concordato preventivo. Una misura simbolo con la quale il Governo ambiva ad ottenere l'impossibile obiettivo di accompagnare con gentilezza e con un sorriso verso la fedeltà fiscale i contribuenti infedeli e recuperare quelle risorse che servono per l'attuazione della restante parte della delega. Ma si è capito presto che questi due obiettivi non sono conciliabili, come ci hanno detto anche i professionisti del settore, i commercialisti e i tributaristi. Infatti i contribuenti infedeli non sono sembrati attratti dal concordato, anche perché contemporaneamente il Governo attuava, con decreti legislativi, misure di allentamento al contrasto all'evasione fiscale, attraverso l'indebolimento di sanzioni e pene e la revisione del sistema giudiziario in materia di questioni tributarie; mentre quelli che già pagano fedelmente le tasse non trovano vantaggio ad aderire a questo strumento. È questa la ragione per cui in corsa, avvisato con *alert* importanti dai dai professionisti, il Governo è dovuto correre ai ripari, provando a rendere ancora più attrattivo questo strumento e introducendo l'improbabile principio della *flat tax* a scaglioni per i redditi eccedenti dichiarati da chi aderisce al concordato. Soltanto in autunno potremo sapere se questa spericolata operazione avrà dei risultati oppure se si tratterà del fallimento definitivo di una misura simbolo della delega. Peraltro - e veniamo alla discussione di oggi - non era molto difficile un anno fa prevedere che oggi ci saremmo trovati a dover prorogare i termini per l'adozione dei testi unici. Una delle contraddizioni della delega - e noi l'avevamo indicato lo scorso anno in discussione - è che essa conteneva due termini diversi per la sua attuazione: come è noto, prevede ventiquattro mesi per i decreti legislativi di attuazione della delega e soltanto un anno per l'implementazione e la revisione dei testi unici. Come può essere possibile che dei testi unici, che possono essere riordinati soltanto a valle di un processo di riforma complessivo,

e più pulito il sistema legislativo, e contro l'essere più chiari rispetto ai contribuenti e ai cittadini. Ma ciò avviene, con buon senso, soltanto dopo che il processo di riforma è avvenuto. Quindi oggi ci troviamo a discutere e a votare su una proroga termini che deriva semplicemente da un errore di valutazione e di prospettiva che il Governo ha commesso un anno fa. Questa è la ragione per cui voteremo contro la proroga dei termini, non potendo però tacere che questi testi unici conterranno revisioni e previsioni legislative che permangono profondamente inique e sbagliate, che assecondano e occhieggiano all'evasione fiscale e che sono in palese contrasto con un principio di equità orizzontale che è nostro dovere costituzionale difendere.

di offesa e di toni alti. Lo dico al collega Turco - per il suo tramite, Presidente - per la stima che porto alla sua competenza e al contributo che dà in Commissione. Parlare

A saldo del tema del fascismo che oggi perlomeno non avete citato, penso che possiamo rassicurare, in questo quadro complessivo di una stagione di riforma, gli italiani, chi ci guarda dall'estero, soprattutto l'Europa, che in Italia non c'è un problema di libertà democratiche. un problema di libertà democratiche. Rispetto al tema che si sta dibattendo della libertà di stampa, credo che una riforma questo Governo debba metterla in campo per quanto riguarda il sostegno alla stampa e per pagare di più i giornalisti. per evitare, come abbiamo sentito in alcuni commenti anche in queste settimane, che qualcuno vada ad abbeverarsi in qualche ambasciata estera e quindi possa dare un contributo non coerente. Penso che nessuno di noi debba essere

alla grande dalla relatrice Tubetti in Commissione, il Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023. a questa stagione di riforme - e lo dico anche con rispetto a chi è alternativo alla nostra visione delle cose e del mondo, a chi vorrebbe tornare ad essere maggioranza

mettesse mano, rispetto ad un'organizzazione orizzontale e verticale dello Stato, a diverse riforme: da quella sul premierato per dare stabilità di Governo a quella sull'autonomia, su cui raccogliete le firme. Per quanto ci riguarda, rispetto a quello che in termini di debito pubblico produce quella parte dell'organizzazione dello Stato locale per noi significa invece responsabilità

viste le grandi riforme. Concordo anche con l'idea che il Parlamento debba tornare ad avere meno decretazione d'urgenza, ma è ovvio che un Governo politico, in ritardo rispetto a quelli che sono gli obiettivi di un'Italia che ricomincia a correre, di un'Italia che ricomincia ad avere fiducia in famiglie ed imprese, aveva la necessità di dimostrare coerenza, affidabilità e quindi anche velocità su tutte queste riforme. Non ultima è quella della giustizia, che ha rappresentato una pietra miliare di questo nuovo patto con i cittadini che, per quanto ci riguarda, restano sempre le famiglie e le imprese. Nella gestione finanziaria 2023, proprio perché i fatti sono chiari, noi riscontriamo che ancora non è intervenuta una riforma fiscale. fiscale. Voglio ricordare che l'Italia è uno dei pochi Paesi europei che non ha codici unici sul piano tributario. Il che significa, rispetto a chi ci guarda dal lato domestico e anche degli investitori esteri, avere grandi preoccupazioni di certezza del diritto, per quanto riguarda gli investimenti e per quanto riguarda anche diritti ed eventuali sanzioni che accompagnano aziende, famiglie e imprese che non sono cittadini operosi dal punto di vista della fiscalità. Quindi, la gestione 2023 ha portato carta canta - anche rispetto al 2022, un aumento di accertamenti in entrata pari al 9,3 per cento: 95 miliardi in più rispetto al 2022. denota un totale di entrate pari a 740 miliardi di euro, quindi con un più 4,2, che sono i 30 miliardi che ci troviamo in più su una previsione di 672; quindi un più 10 Tutte maggiori entrate tributarie di quel Governo, annunciate da Tele Meloni, con lo spauracchio che doveva portare a grande evasione, a grande sfiducia, a non avere la tenuta sociale economica. Voglio ricordare, anche rispetto alla memoria di questo confronto, di questo benchmark con gli altri Paesi europei, che quest'Italia forte solida vale anche rispetto a quella popolazione dell'Emilia-Romagna, che è un po' più avanti della classe

già annuncio, prima della fine del mio intervento, il voto favorevole del partito che ancora oggi ha la fiducia e la maggioranza degli italiani, perché anche su quello c'è un principio di lealtà alla nostra convivenza sociale e civile. *(Applausi)*. Voglio ricordare a me stesso, in un esercizio che non deve essere retorico, come funziona la nostra tenuta per far sì che non succeda da noi quello che è accaduto in Spagna, in Argentina, in Grecia, anche con speculazioni voglio ricordare ai costituzionalisti da Bignami che fare le leggi di bilancio in questa stagione politica è molto più complesso. Lo avete provato anche voi, però, sulla vostra pelle, anche se erano Governi eterogenei, che non reggevano. Quindi, vale anche anche per il nostro collega Renzi, cui guardiamo con grande simpatia, che ormai continua a dare consigli non richiesti, una volta a destra e molto a sinistra. Meno male, insomma, che cominciano a non accettarli dato che il suo grado di affidabilità, anche nei confronti degli italiani, si è già abbastanza ridotto.

cento) passa da 50 miliardi a 57,5 miliardi. Anche l'IVA ha sull'accertato un 2,2, ossia 4 miliardi in più. Questo testimonia che,

il cosiddetto redditometro, che era uno "spiometro", in una "evasometro". Il che significa andare a rintracciare con gli strumenti di intelligenza artificiale il grande lavoro dell'Agenzia delle entrate e, quindi, la riscossione e l'adesione ideale a un'Italia che rialza la testa, che è quello che ci testimoniano famiglie e imprese. Voglio ricordare anche in queste ultime ore i nostri atleti alle Olimpiadi, perché in quella stoccata di chi utilizzava la spada c'erano la soddisfazione e il *sentiment* di un Paese che rialza la testa. La differenza sta proprio qui: di immaginare che queste riforme accompagneranno stagioni che riguardano le nostre famiglie e le nostre imprese. Ci sono tre formule: una è quella dell'austerità, che noi abbiamo combattuto non soltanto sul piano non solo ideologico, ma anche politico. In Europa la Meloni è stata coerente rispetto a un'accozzaglia di numeri che creano maggioranze per occupare poltrone occupare poltrone e sono quelle, ad esempio, che vorrebbero stratassare la casa degli italiani, che insieme ai nostri risparmi rappresenta un bene su cui il 70-80 per cento degli italiani ha messo le proprie risorse. Per cui non ci restava che organizzare meglio lo Stato; combattere l'evasione e avere gli introiti che stanno già arrivando; evidenziare con riforme complessive - e questo è un pezzo di tutte quelle riforme che in questi provvedimenti d'urgenza si stanno discutendo nei due rami del Parlamento quella che è l'azione di un Governo coraggioso. Mi pare di poter dire ai miei colleghi della maggioranza che occorre rivolgere un grande plauso, a dispetto di una sottovalutazione che è anti-italiana, al grande lavoro del ministro Giorgetti e del vice ministro Leo, per quello che stanno facendo, rispetto alla considerazione internazionale e rispetto a una

segnalare a quest'Aula, all'attenzione dei colleghi e - se qualcuno lo riporterà - al Ministro della salute, un ennesimo caso che si potrebbe definire di malasanità, ma che secondo me dà il segno di quanto siano in sofferenza anche gli operatori sanitari che si trovano ad affrontare, in carenza di organico, le esigenze quotidiane dei cittadini italiani nei nostri ospedali. Come riporta un noto quotidiano torinese, qualche giorno fa un un cittadino ha accompagnato la madre al pronto soccorso per un dolore al petto in orario serale. L'anziana donna, di ottantasette anni, è stata trattenuta in osservazione durante la notte. Il figlio si era raccomandato di chiamarlo all'indomani in caso di dimissioni; sennonché nessuno ha contattato il familiare e la donna è stata trovata vagare alle ore 11 del mattino successivo nei successivo nei pressi di casa, in cerca della propria dimora. Ovviamente il figlio, informato da una vicina, è accorso a prendersi cura della madre - ripeto ha fatto delle rimostranze nei confronti del personale sanitario dell'ospedale dov'era stata ricoverata durante la notte. Non vi leggo le risposte che possono sembrare un un po' surreali di chi ovviamente aveva di fronte un cittadino scontento delle prestazioni erogate o quantomeno dell'esito del mattino dopo. Ecco, quando parliamo di personale che è esaurito, che non sa come affrontare ogni giorno il sovraccarico di lavoro, mettiamoci nei suoi panni: magari la signora sembrava attenta e alla domanda se sapeva tornare a casa, avrà risposto di sì e quel personale, preso da mille incombenze, non ha pensato a chiamare il familiare. Avere poco personale nei nostri pronto soccorso vuol dire anche questo. Quindi, quando noi chiediamo di assumere personale e di prestare attenzione alla nostra sanità, è perché esistono anche questi problemi. Questo non è un reale caso di malasanità, perché per fortuna la signora sta bene, ma sicuramente le cose potevano finire decisamente peggio e avremmo potuto leggere quest'oggi sui giornali di un'anziana trovata in chissà quale condizione e chissà dove, perché dimessa senza attenzione da uno dei nostri pronto soccorso. Oltretutto segnalo che si tratta di un pronto soccorso di un'eccellenza torinese, uno di quegli ospedali dove uno pensa di essere fortunato se mandato lì con un'ambulanza. Quindi, figuratevi quando vi mandano in quelli in cui vi ritenete già sfortunati solo a sentirne il nome. Ecco, quando diciamo che la nostra sanità va finanziata meglio, è anche per questi motivi.

Grazie Presidente, domani mattina alle ore 12,20, una ragazza italiana, una ragazza della provincia di Napoli, di Afragola, salirà su un *ring* alle Olimpiadi e andrà a combattere la sua battaglia, dopo anni dedicati alla boxe, contro un trans. Io trovo che questa sia una cosa che debba far riflettere perché, per la prima volta in mondovisione, un uomo picchierà una donna.

una ragazza italiana della Polizia di Stato, delle Fiamme Oro, sarà presa a pugni da una persona in base al percepito, e non in base a ciò che è.

passa il percepito. Qualsiasi discriminazione va combattuta, nei confronti dei trans, nei confronti degli omosessuali, ma anche e soprattutto nei confronti delle donne che, con il precedente di domani, avranno diritto a meno medaglie *(Applausi),* avranno diritto a prendere i pugni in faccia e nessuno dice niente, né le femministe, né le tante donne di centrosinistra che adesso stanno urlando e si dovrebbero vergognare. *(Applausi)*. Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea un fatto grave che, se confermato - proprio come accennava il collega - si dovrebbe consumare domani sul ring della boxe femminile alle Olimpiadi di Parigi. Le sue ripercussioni, se confermate, si abbatterebbero come uno tsunami su anni di orgogliose battaglie e legittime rivendicazioni delle donne di potersi affermare anche nel mondo dello sport. È noto, infatti, che alle Olimpiadi, domani la nostra pugile azzurra Angela Carini, dovrà incontrare sul ring non un'altra donna, ma - da quello che leggiamo sulla stampa nelle ultime ore - un uomo che, per mezzo della transizione, oggi è stato ammesso a combattere contro le donne. Se confermato, ci troveremmo di fronte a un uomo che combatte contro le donne. Dovevano essere le Olimpiadi della parità raggiunta, almeno numericamente, fra gli atleti uomini e le atlete donne in competizione; un 50 per cento voluto e perseguito che, se paragonato al 4,4

invece di essere ricordate per essere quelle della slealtà competitiva, dei passi indietro per l'affermazione femminile; quelle che legittimano nuove forme di sopraffazione verso le donne, costrette a combattere con chi invece ha una struttura fisica e la forza di un uomo. Oggi ce ne accorgiamo perché ad essere coinvolta è un'atleta italiana, ma questo non è il primo caso in cui si parla di disparità, o meglio di ingiustizia, dovuta a caratteristiche biologiche che si registrano nel mondo dello sport. È il caso di Terry Miller e Andraya Yearwood che sono delle *sprinter* del Connecticut, che si identificano come donne e dal 2017 partecipano e vincono tutti i più importanti campionati scolastici e statali di atletica, lasciando indietro le coetanee, stabilendo nuovi *record* e soffiando loro trofei e medaglie. Questo è stato sottolineato anche da atlete donne come Martina Navratilova, paladina dei diritti LGBT, che ha dichiarato esplicitamente non essere giusto e onesto che le donne gareggino, ad esempio, contro la *transgender* Lia Thomas. Da Vice Presidente della Commissione bicamerale sul femminicidio e ogni altra forma di violenza contro le donne, voglio dire che tutto questo non può e non deve diventare una nuova normalità. Non può e non deve essere accettato in nome di una presunta inclusione ciò che in realtà si può trasformare in una discriminazione contro le donne. Per chi difende le donne questo non è il tempo del silenzio. Le donne non si toccano neppure con un fiore, recita un noto detto; eppure non sembra corrispondere a ciò che l'ideologia woke potrebbe quotidianamente portare avanti e domani consumarsi su quel ring. Noi siamo qui per questo, per difendere le donne, e a tutte quelle atlete, come la nostra Angela Carini, che per anni si allenano per arrivare alla competizione forse più ambita della loro carriera sportiva, pochi giorni a disposizione per raccogliere i frutti di anni di lavoro e di sacrifici, noi diciamo che noi siamo e saremo lì a difenderle.

vorrei segnalare una serie di inesattezze che oggi il ministro Salvini, in risposta a un *question time* alla Camera, avrebbe detto in riferimento all'assegnazione degli alloggi popolari da parte del Comune Che cosa è successo? Siccome sono stati assegnati degli alloggi ad alcuni degli abitanti del campo rom di via Bonfadini, Bonfadini, recentemente sgombrato proprio dall'amministrazione di centro sinistra, il ministro Salvini, rispondendo ad un'interrogazione di alcuni membri della maggioranza, avrebbe detto che questa è una scelta discrezionale del Comune di Milano e, quindi, si era dimostrato molto preoccupato. preoccupato. Vorremmo ricordare al ministro Salvini, che ha anche la competenza per quanto riguarda il tema dell'abitare e quindi dovrebbe occuparsene, che non si tratta di una scelta discrezionale del Comune di Milano, ma sostanzialmente gli alloggi SAT sono delle soluzioni abitative transitorie che il Comune può assegnare in condizioni di fragilità accertata, in aggiunta agli alloggi previsti dal piano annuale, secondo quanto previsto da una legge varata dalla Regione Lombardia a tutela delle fasce deboli in stato di necessità. Infatti, non è un caso andrebbe sottolineato che questo strumento sia stato usato proprio dalla Regione guidata dal presidente Fontana nel novembre del 2022, per lo sgombero delle case ALER di via Bolla.

e che quindi decide insieme in che modo poter assegnare alloggi, secondo una legge regionale, in situazioni di grave ed estrema difficoltà. difficoltà. Penso che evidentemente il Ministro non fosse informato e questo già lo ritengo grave, perché in tal caso non conoscerebbe una legge della Regione Lombardia e soprattutto come stanno le cose. come stanno le cose. Se invece il Ministro avesse per caso mentito e raccontato una storia nello *storytelling* delle *fake news* per gettare benzina sul fuoco, questo sarebbe ancora più grave.

Che gli piaccia o no, quest'Aula è fatta per confrontarsi, e se può smentire anche solo una delle mie affermazioni riguardo al provvedimento o all'operato del Governo, lo Grazie, si faccia una domanda. Ribadisco che, se il senatore Sigismondi può smentire anche solo una delle mie affermazioni, può farlo qui in quest'Aula, altrimenti si rassegni al triste ruolo di comparsa. *(Applausi)*.

Grazie,